quantomeno sconvocare le Commissioni e riconvocarle in un orario in cui il nostro Gruppo possa essere presente, perché diversamente ci diventa impossibile svolgere il nostro lavoro.

autonomia. Credo che la cosa migliore da fare sia interloquire con le Presidenze delle due Commissioni e far presente il problema. Successivamente sono sono convocate le medesime Commissioni per affrontare altri argomenti e quindi potrebbe essere utilizzato l'orario già stabilito.

la stessa definizione contenuta nel decreto‑legge, in modo particolare all'articolo 9. Signor Presidente, vorrei altresì illustrare l'emendamento l'emendamento 1.37, riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

sotto i 15.000 abitanti. In primo luogo, ci sembra assolutamente assurdo che i Comuni virtuosi, che hanno una grande capacità dovuta alla loro volontà di lavorare, garantendo i servizi con le poche risorse che gli rimangono,

locale. Chiediamo che ci sia la volontà del Governo di aprire in questo senso, superando il pareggio di bilancio, per dare risposte concrete che vanno poi a toccare risorse già esistenti nei piccoli Comuni.

In Commissione è stato svolto un grande lavoro sugli emendamenti, perché erano pochi e quindi li abbiamo potuti esaminare bene. In quella sede ci si è accordati sostanzialmente sulle riformulazioni

poche parole sull'emendamento 1.37, illustrato dalla senatrice Comaroli. Mi spiace, ma debbo insistere. Come ho già detto in Commissione,

già oggi non è oggetto di impegno. Quindi, se noi scrivessimo in questa norma e accettassimo il fatto che c'è bisogno di un emendamento per chiarire questo punto (che riguarda il fatto che, non essendo oggetto di impegno,

cui parlo si sono trovati in una condizione di difficoltà e, quindi, di sforamento in ragione di ritardi nel trasferimento dei fondi regionali.

merito non si intacca minimamente la finanza dello Stato, perché stiamo parlando di risorse che sono comunque nella disponibilità degli enti locali e che derivano direttamente dal bilancio della Regione.

Signor Presidente, non ripeto quanto già detto sull'articolo 1. Anche sull'articolo 2 i pareri agli emendamenti presentati sono tutti contrari.

il Governo ha deciso i nuovi LEA che le Regioni devono prestare ai cittadini.

per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo emendamento, che indubbiamente è opportuno. Per poter lavorare sul bilancio,

che si occupi di quest'area, relativo al fatto che i Servizi del bilancio del Senato e della Camera dovrebbero poter avere la stessa possibilità. È evidente che, se non ha se non ha questa possibilità il Parlamento, sarebbe davvero bizzarro che altri possano averla, ma non la Camera e il Senato. Quindi, nel dichiarare il voto favorevole, auspico che in un futuro si affronti anche la questione dell'accesso a quei dati da parte dei Servizi

su quanto deciso ieri dalla Conferenza dei Capigruppo, insieme a lei, Presidente, nel richiedere al Governo (presente in quel momento il sottosegretario Pizzetti)

una serie di motivi che è facile comprendere. Vale a dire, se noi non riusciremo a rimettere in discussione quella procedura del *bail in*, come mi pare da più parti richiediamo senza che poi il Governo riesca a rappresentarlo in sede europea, non so quali saranno i risparmiatori che verranno tutelati così come dice sui giornali il ministro Padoan. Il Ministro si riferisce ai risparmiatori del Monte dei Paschi di Siena o si riferisce ai risparmiatori italiani? Perché, ad esempio, come leggiamo e come già accaduto con la partecipazione al fondo Atlante, la Cassa depositi e prestiti dovrebbe essere impegnata in un'operazione di garanzia su una gigantesca situazione di sofferenze; gigantesca a seconda dei punti di vista, perché se valutiamo gigantesche le sofferenze delle banche italiane, come dovremmo valutare allora gli effetti, ancor più che giganteschi, del peso dei derivati sulle banche, non solo italiane ma soprattutto tedesche, il punto è un altro, signor Presidente, e lo esprimo molto rapidamente Il nostro ministro Padoan, impegnato in questa trattativa che penso sia quasi del tutto conclusa, ma che vorremmo fosse oggetto anche della conoscenza e dell'informazione del Parlamento e non solo dei giornali, immagino che ieri debba aver provato molto imbarazzo durante la riunione dei Ministri economici, quando il suo omologo ceco - ma che ci sente benissimo - ha definito la situazione delle banche italiane peggiore della Brexit, dal punto di vista degli effetti della ricaduta sul sistema europeo e quindi anche sul nostro Paese. Non ho compreso bene, perché non ci non ci vedo e non ci sento bene come il ministro Babis, se egli si riferisse al fatto che anche le banche italiane dovrebbero uscire dall'Europa come ha fatto la Gran Bretagna e quindi poter continuare ad esistere come banche in virtù di questa perché dentro questo sistema di regole europee le banche italiane sono la vittima predestinata di una grande speculazione internazionale, che si sta abbattendo ancora una volta sul nostro Paese.

di stare dentro un contesto in cui gli unici a essere penalizzati siamo sempre noi. È di questo che ci deve informare il ministro Padoan; deve cioè informare l'unica sede della rappresentanza dei cittadini,

se non con le parole di circostanza che egli (molto ben educato) ha utilizzato, ma che non rendono l'idea di come l'Italia si dovrebbe difendere, signor Presidente del Senato, da un attacco gravissimo ai risparmiatori italiani. Questo, infatti, non è l'attacco alle banche ma ai ai risparmiatori italiani; è come portarci via quel poco che ci resta chiedendoci di rispettare regole che non abbiamo mai condiviso, che un Parlamento distratto ha votato in una giornata di luglio un anno fa, senza capire che stava mettendo

proverò a farlo io e mi auguro che lo faccia il Parlamento intero, quantomeno le forze di opposizione. Ricordo al Ministro delle finanze di uno staterello abituato a fare bicchieri di cristallo un grande Paese, fondatore di quest'Europa, con un sistema economico che non ho bisogno di raccontare né in questa sede né al ministro Babis, un signore che faceva la spia per i servizi segreti russi, che si è trasformato in un magnate dell'agroalimentare e che oggi si permette di dare lezioni di liberaldemocrazia - come dice lui - in quest'Europa e al mio Paese. A lui io rispondo che è liberaldemocratico come io sono la regina Elisabetta e siccome non sono la regina Elisabetta, lui con la liberaldemocrazia non c'entra niente. Pretendo però che il Governo del mio Paese, mai eletto dagli italiani ma che ha la fiducia di questo Parlamento, difenda la dignità e la forza del nostro Paese e l'onore dei nostri risparmiatori, della gente italiana che ha risparmiato, costruito quest'economia e che questo Governo rischia di mandare a rotoli. Io pretendo che il ministro Padoan venga in Aula

italiano è sotto attacco della finanza speculativa, ma è anche vero che nell'ultimo anno questo Parlamento si era impegnato a istituire una Commissione d'inchiesta per arrivare a individuare le responsabilità del sistema bancario italiano e quali siano i soggetti

quello che il Parlamento ha deciso e non quello che lui vuole fare. Ricordo infatti quello che è stato fatto nell'ultimo anno da questo Governo al sistema bancario italiano e ai risparmiatori, che devono essere e tutelati e non truffati, come è successo. sede e riportare la voce del Parlamento, che per ora è l'unico sovrano, perché *mister* Renzi non è assolutamente sovrano e non è in grado di gestire questa difficoltà

Penso che la saggezza di quest'Assemblea aiuterebbe anche lui a confrontarsi con tematiche che non ci sembrano marginali in questo momento. È vero, in fondo, che non ci si può permettere di accettare le accuse di un Ministro di un altro Paese che parla delle nostre banche; ma è anche vero che finché il

essere interpretato al mattino leggendo i giornali; forse un po' di rispetto anche per questo Parlamento sarebbe utile per rafforzare le posizioni dell'Italia in un contesto difficile. Magari Magari sarebbe meglio avere più rispetto per il Parlamento che per certi banchieri che, come si è visto oggi sui giornali, sono riusciti ad aumentarsi gli stipendi del 9,7 per cento in quest'ultimo anno, nonostante l'ampia responsabilità che hanno a tutti i livelli, anti-*crack*. *(Applausi del Gruppo LN-Aut)*. Signor Presidente, penso che tutti noi, a prescindere dal colore politico, rappresentiamo qualcosa e qualcuno e lo rappresentiamo con la lealtà verso i nostri elettori. Il Governo non è stato eletto ma in questa sede trova la fiducia di una maggioranza: venga a riferirci la verità sulle

anche Forza Italia si associa alla richiesta che il ministro Padoan venga a riferire in Aula. Vorrei sottolineare che credo sia nell'interesse del Paese

che gli eventuali problemi di una banca si riversassero sul contribuente. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che quando interviene lo Stato significa che intervengono i contribuenti italiani: i soldi non arrivano dal cielo, ma dai contribuenti. Era teoricamente giusto che non fossero addossati alla collettività gli errori dei dirigenti delle banche che andassero in difficoltà. Ma lo stesso *bail in* prevede che, in casi straordinari, ci possano essere delle eccezioni. Ora, il perdurare della crisi economica che attanaglia tutta l'Europa

conciso ma serio e meditato, alla fine si potrebbero approvare delle risoluzioni in grado di dare la forza al Governo di presentarsi

i cittadini e i risparmiatori sono senza alcun tipo di informazione e rischiano, visti i precedenti, di vedere tutti i loro sacrifici e i loro risparmi

In primo luogo, in sede europea numerosi e autorevoli esponenti danno per scontato il ricorso al cosiddetto fondo salva Stati da parte del Governo italiano

visto che il Presidente del Consiglio italiano ha più volte reiterato l'invito ai nostri risparmiatori a stare sereni. Il secondo fattore è ancora più complesso. Da qualche giorno c'è uno scambio di "effusioni" tra il Presidente del Consiglio in carica e un ex Presidente del Consiglio, anch'egli facente parte del Partito Democratico, che altro non sono che vere e proprie notizie di reato.

alle intese internazionali sia in relazione agli incontri che stanno avvenendo sul suolo patrio. Riconfermo questa disponibilità. Ciò detto, vorrei dire con nettezza che questa polemica sul Governo e sul *Premier* non eletti è abbastanza stucchevole, tanto più che siamo in una Repubblica parlamentare e la fiducia ad un Governo in una democrazia parlamentare la dà un Parlamento. Questo Parlamento ha dato la fiducia al *Premier* e al Governo.

a maggiore ragione, dovrebbe essere loro chiaro lo stato dell'arte di una Repubblica parlamentare. Rispetto naturalmente lo spirito nazionale e di difesa degli interessi nazionali, che ho sentito evocare a difesa, appunto, degli interessi dell'Italia e dei risparmiatori italiani. Penso che il Governo su questo sia alacremente impegnato e non condivido le parole che sono state riservate ad un esponente di un Governo europeo, che naturalmente rimangono nella responsabilità di chi le ha espresse,

dal senatore Vacciano». Il senatore Vacciano, con lettera del 12 maggio scorso, ha reiterato le proprie dimissioni, già respinte nelle sedute del 17 febbraio e del 16 settembre 2015.

ma perché credo davvero che nel corso delle altre due discussioni sia stato detto tutto o almeno tutto ciò che poteva essere necessario per far comprendere la natura e la piena libertà della scelta da me fatta. Al collega Buemi, che rimarcava la natura politica del mio gesto, non posso che confermare tale interpretazione. Ribadisco che, per quanto mi riguarda, questo non dovrebbe essere un ostacolo, ma al contrario la scelta più coerente e rispettosa della volontà espressa da coloro i quali continuo a considerare i miei datori di lavoro: i cittadini. Perché, nella mia modestissima esperienza da portavoce, questo è la politica: servizio civile e rispetto dei cittadini. Quei cittadini che tramite una legge incostituzionale hanno solo potuto decidere di affidare il proprio voto ad anonimi volti dietro un simbolo. Vedete, colleghi, il fatto che non mi riconosca più in quel simbolo e il giudizio che ho delle sue attuali dinamiche sono assolutamente ininfluenti. Il giudizio sull'operato e sulle dinamiche del Movimento 5 Stelle lo esprimeranno gli elettori alle prossime politiche: al momento ci sono 9 milioni di persone che hanno diritto ad un portavoce in più in Senato e che meritano esattamente lo stesso rispetto che va tributato a questa istituzione. È con loro, non con simboli o capi di partito, che ho preso il mio impegno. Ringrazio i colleghi che hanno avuto parole cortesi, lusinghiere e probabilmente immeritate nei miei confronti e in particolare il senatore Falanga, con il quale ho avuto un breve confronto dopo il voto scorso. Tuttavia la politica, per come l'ho vissuta, necessita di qualcos'altro oltre all'impegno, alla preparazione e allo studio; necessita di amore e di passione e io quell'amore e quella passione, semplicemente, non li ho più, perché erano legati a doppio filo con la mia esperienza nel Movimento 5 Stelle. Rimane il senso del dovere di chi, con tutti i limiti del caso, cerca di svolgere al meglio la mansione affidatagli perché, come già detto, nutre grande rispetto nei confronti del proprio "datore di lavoro". Con molta umiltà, credo che questo Paese meriti di più. Presidente, colleghi, le mie idee sono molto distanti da quelle della maggior parte di voi, ma è stato un onore avere la possibilità di confrontare quelle idee e quindi, nel concludere rinnovando la richiesta di accoglimento delle mie dimissioni, auguro con sincerità buon lavoro a tutti voi e un grande in bocca al lupo agli italiani.

nel 2012, quando con i miei colleghi ci siamo candidati in Parlamento sotto l'egida del Movimento 5 Stelle, eravamo mossi convintamente dalla volontà di cambiamento. Come i nostri elettori, vedevamo nel Movimento 5 Stelle la legittima difesa del popolo italiano. Siamo entrati nelle Aule di Camera e Senato lasciando in *standby* le nostre carriere professionali, per chi ne aveva una, e in certi casi anche rimettendoci economicamente e in salute. All'inizio eravamo del tutto ignari del funzionamento della macchina, dal *drafting* legislativo ai rimborsi. I rimborsi, quelli che il Movimento 5 Stelle continua a dire di non prendere e che noi invece sappiamo benissimo vengono usufruiti in modo anche leggero per quanto riguarda i Gruppi. I rimborsi vengono fuori dappertutto e sono male amministrati, a beneficio di fedelissimi che continuano ad attingere senza rispettare le esigenze di tutti. Sono quindi venute meno quella coralità e quell'alta politica che volevamo cambiare. Oggi ci troviamo a discutere l'ennesima richiesta di dimissioni del senatore Vacciano, deluso dalle malefatte interne del Movimento, di cui convintamente facevamo parte,

Egli se ne andò per protesta dopo la nomina dall'alto, in blocco, dei ragazzotti del cosiddetto direttorio. Ora abbiamo un futuro

con ciò che la comunicazione gli fa recitare a *slogan* e rigorosamente riassunto a titoli. Ebbene, questo non è il Movimento 5 stelle per cui Vacciano si è candidato allora e non corrisponde nemmeno al mio Movimento 5 Stelle. Il nostro Movimento non prevedeva tanta ipocrisia e non comprendeva tanto oscurantismo, tanta mancanza di trasparenza, tanta scorrettezza Non generalizzo, perché nel Gruppo ci sono delle persone che stimo profondamente, ma il sistema e l'andazzo prevalenti che sono emersi esulano da quella buona politica di cui ci siamo innamorati. La politica è un po' così, viene un po' per passione - la politica è passione - e ci siamo ritrovati tutti coinvolti forse anche un po' casualmente. Io sono per una politica che deve essere alta, cioè una politica del fare, ovvero di governare la città e chi la abita (cioè la società)

Una buona politica deve soddisfare le richieste dei cittadini, è coerente con le intenzioni, si rende comprensibile e ha in se stessa gli strumenti per correggersi e cambiare in meglio: buona politica che deve prendere origine dal senso originario di amministrazione della *polis*, ma che deve diventare una politica più alta, una sfera

sotto l'egida dello sgomitamento e della prepotenza di alcuni, ma in una vera e propria oclocrazia. In questo contesto, la presenza del collega Vacciano in questo Parlamento (lui, persona perbene, esperta in finanza, che ha fatto sempre fatto il suo lavoro e che si interroga sull'opportunità o meno di restare)

non sei tu a esserti distaccato dal Movimento, ma è il sogno del Movimento che, con l'addivenire, è diventato qualcos'altro e ha tradito se stesso. Ci sono tanti elettori delusi, come te e come me, che in te invece si riflettono e rispecchiano tuttora. C'è una ragion di Stato che va oltre le esigenze personali, le difficoltà ed anche il peso che ognuno di noi In questi ultimi anni siamo andati purtroppo degenerando sempre più, facendo una politica di *slogan*, di partito visto come azienda. E sembra proprio che ogni volta venga sempre meno il principio democratico di confronto di idee, di campo aperto

che sta qua e che si interroga sull'utilità e sul ruolo che noi tutti veniamo ad assumere. Aggiungo un'altra cosa. Recentemente, tra le varie critiche che sono state fatte a Renzi, Speranza ha detto che non ha guidato il partito, come se questa fosse una nota cattiva, di demerito. Ebbene, io invece penso l'obiettivo non debba essere la salvaguardia di un partito, ma la salvaguardia del bene di uno Stato e di un Paese e di idee che non hanno non hanno partito e maglietta. Per cui il buono di Vacciano e le idee di Vacciano si possono realizzare ed esprimere tutt'oggi, anche sotto un'altra maglia, anche sotto un altro simbolo, anche sotto nessun simbolo. Ci tengo che lui ci sia. Nella peggiore delle ipotesi, proporrei una soluzione quasi salomonica di scambio: mi metterei io al posto di Vacciano, però non lo farei gratuitamente: lo potrei fare concordando l'approvazione di due o tre disegni di legge cui tengo particolarmente. Dopodiché me ne potrei andare immediatamente, perché la mia funzione sarebbe compiuta. Mentre molto più coerente ed utile la presenza di Vacciano, che invito a restare, anche con qualche esitazione, e non soltanto ad esserci e a continuare benissimo quello che sta facendo, ma a ritrovare l'entusiasmo e a sentirsi la persona giusta al posto giusto.

fatti. Quando il collega Vacciano fece delle critiche sulla costituzione di questo cosiddetto direttorio, il Gruppo parlamentare si interrogò e ovviamente ne discusse in un'assemblea,

Stavo dicendo che il Gruppo parlamentare si trovò a decidere se continuare a tenere al proprio interno il collega Vacciano. Il Gruppo dei senatori

c'è il Capogruppo di turno che si trova a fare il portavoce della Casaleggio Associati. All'epoca c'era lo stesso Gianroberto Casaleggio, che telefonò al Capogruppo e decise l'espulsione dal Gruppo del senatore Vacciano; e così avvenne. Sinceramente le motivazioni del collega Vacciano (un collega che stimo, perché vedo come svolge correttamente il proprio mandato), non mi hanno convinto. Abbiamo tutti quanti ricevuto un mandato parlamentare e siamo dei rappresentanti. Al momento non sono i cittadini a decidere se dobbiamo continuare o no

è stato scritto dai Padri costituenti; se vogliamo aprire una riflessione, ben venga: discuteremo sulla legge che regolamenterà i partiti; si potrà anche non dico modificarla, ma instaurare un dibattito su come devono essere regolamentati i partiti. Ma attualmente queste cose non sono previste. mi sembra che finora il collega Vacciano abbia continuato e continui a svolgere il proprio mandato partecipando sia ai lavori dell'Assemblea che ai lavori della Commissione. Commissione. Per questi motivi, invito l'Assemblea a riflettere attentamente su questo voto. Non si tratta tanto del fatto di discutere della richiesta delle dimissioni del collega Vacciano, che ovviamente nessuno di noi ha la facoltà di nonostante ci sia un principio nel nostro Regolamento che verrà ripreso, qualora verrà approvata la nuova Costituzione, del dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Un concetto sul quale dobbiamo riflettere riguarda invece il valore di una decisione esterna a un Gruppo parlamentare sulla presenza di un parlamentare all'interno di un Gruppo.

intelligentemente proprio per raggiungere questo obiettivo, perché ricordo le parole del collega Morra quando si insediò come Capogruppo e affermò che voleva avere 52 fratelli, e quant'altro; il giorno dopo arrivò la decisione e con l'amico Crimi firmò l'espulsione della collega Gambaro.

Signor Presidente, aggiungo una mia riflessione, se i colleghi me lo consentono, alla vicenda delle dimissioni del collega e amico senatore Giuseppe Vacciano, persona integerrima, di grande competenza e gran lavoratore. Vede, senatore Vacciano, le sue dimissioni per motivi personali o politici, come lei ci ha illustrato, non sono nella sua disponibilità piena,

Perché è compito di questa Assemblea valutare pienamente se le sue dimissioni sono frutto di pressioni esterne. Io credo, caro collega,

Quei nove milioni di elettori, infatti, non hanno votato un Movimento che, nello spregio totale delle regole, non solo interne, che si è dato, ma anche nello spregio del più banale vivere in una società civile e democratica, ha operato nel senso che ci ha ricordato adesso il senatore Battista. Il Movimento l'ha espulsa senza passare né da una Assemblea parlamentare né da un voto della rete.

nel decidere le sue dimissioni, fattori che esulano dalla sua stessa volontà, per una questione di tutela del suo stesso ruolo. Ebbene, noi non possiamo che prendere atto di quanto accaduto

di un'azienda privata che è riuscita, tramite pressioni, dirette e indirette, a far dimettere un parlamentare della Repubblica.

Per queste motivazioni, signor Presidente, invito tutti i colleghi a prendere la decisione di respingere queste dimissioni, cosa che farò senz'altro anche

alcun principio ma, anzi, siamo proprio di idee contrapposte. Ma è questo il seme e l'essenza della democrazia. Questo è il vero dibattito democratico. Tu stesso hai detto, collega Vacciano, che hai idee completamente diverse da molti di noi. Ma è proprio il confronto tra le idee che fa andare avanti la democrazia. I nostri Padri costituenti, da La Malfa, a Pertini, a Calamandrei, a De Gasperi, a Saragat, a Terracini, a Malagodi (per citare tutti quelli dell'arco costituzionale della Prima Repubblica), hanno inteso proprio questo.

che si contrappone alla nostra. E questo dibattito noi lo vogliamo continuare, perché è questa la democrazia. Io non conosco le pressioni delle

Signor Presidente, rispetto molto il punto di vista del collega che ripropone a quest'Assemblea le sue dimissioni,

provvedimento sui partiti democratici dovrebbe impedire che avvenga nel nostro Parlamento quello che sta accadendo.

ma abbiamo un dovere prioritario e fondamentale che è rispondere prima di tutto alla nostra coscienza e ai nostri principi, quelli scritti in Costituzione e quelli che pensiamo di avere condiviso nel momento in cui ci siamo candidati, che siano rappresentati dal Movimento 5 Stelle o dal Partito Socialista Italiano. Noi abbiamo quest'obbligo e non non può venir meno, né perché qualcuno tende a buttarci fuori, né perché non riteniamo più possibile stare dentro. Siamo un'entità protetta dalla nostra Costituzione nelle nostre posizioni politiche, che sono, appunto, espressione dell'esercizio della funzione parlamentare senza vincolo di mandato. Dal momento in cui entriamo qui dentro, a prescindere se siamo eletti dai piemontesi o dai siciliani, dal Partito Socialista o dal Movimento 5 Stelle, rispondiamo prima di tutto alla nostra coscienza e al nostro ruolo principale che è quello di interpretare il momento storico, gli interessi generali del Paese o gli interessi di quei settori che intendiamo rappresentare in questa sede. Se vogliamo svolgere fino in fondo questo mandato non possiamo arrenderci, caro collega, non possiamo battere in ritirata. Ammetto solo due ragioni per l'abbandono: il grave stato di salute e gravi misure giudiziarie. Il resto è un abbandono, un tradimento al mandato principale ricevuto.

le sue dimissioni dal Senato. Vorremmo ricordare come la nostra Costituzione dia centralità alla persona, all'eletto, e non ai partiti. La Costituzione ha sempre difeso l'eletto e la libertà dell'eletto. Le immunità e le garanzie servono al parlamentare per esercitare appieno il mandato. In primo luogo, servono garanzie perché si possa discutere senza aver paura di essere incriminati; in secondo luogo, servono garanzie anche per proteggere dalle pressioni dei partiti, perché la libertà sia verso l'esterno ma anche verso l'interno. Questo dice la nostra Costituzione e questo dicono i sistemi democratici. L'alternativa è la dissoluzione parlamentare:

è il singolo e la libertà del singolo; in alternativa, nove persone, con voto ponderato, alzano le mani: uno conta per 113 voti,

Signor Presidente, intervengo a titolo personale in questa discussione, senza far riferimento alle vicende che riguardano gli ex e gli ancora presenti nel Movimento 5 Stelle, tengo a testimoniare come, dall'osservatorio privilegiato della Commissione finanze, di cui anche il senatore Vacciano fa parte, ho potuto conoscere ed apprezzare le qualità del nostro collega. Voglio citare in particolare la competenza e la serietà con cui affronta le questioni, a volte anche molto tecniche, con cui la Commissione si confronta, la tenacia con cui approfondisce i temi e sostiene il proprio punto di vista, accompagnato però da una disponibilità vera

difficile compito di soppesare, da una parte, la correttezza di assecondare la richiesta che ci viene oggi ripresentata dal senatore Vacciano, nel rispetto della serietà della persona che la rivolge (e questo è un punto che sottolineerei con forza e che mi sembra sia stato

e quindi la collettività di un contributo di rilievo che abbiamo imparato ad apprezzare. Nel segreto del voto ciascuno dovrà fare la scelta tra questi due elementi, entrambi importanti.

mediante procedimento elettronico sulle dimissioni reiterate dal senatore Vacciano. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo oggi in discussione modifica la legge n. 243 del 2012 intervenendo sul tema degli equilibri dei bilanci di Regioni ed enti locali. Mi auguro, sia da senatore della Repubblica che da presidente di ANCI Puglia, che tale modifica possa fare definitivamente chiarezza sul punto in questione, nonostante alcuni nodi irrisolti che qui illustrerò. Come sapete, nell'ottica del superamento del Patto di stabilità interno, i bilanci degli enti locali dal 2009 sono stati al centro di sperimentazioni e modifiche normative. Forse troppe! Ciò non toglie, come anticipavo, che un commento critico a questo disegno di legge si possa e si debba fare. Permettetemi, dunque, alcune riflessioni e alcuni passaggi tecnici. Per prima cosa voglio ricordare due osservazioni della Corte dei conti che ha sottolineato che questa norma ha alcune contraddizioni perché non si adatta ai criteri sull'attuazione del pareggio di bilancio. In tale modo, detto più semplicemente, produce l'ennesimo mancato coordinamento con altre due normative precedenti. Siamo purtroppo ad un antico difetto italiano: sempre più leggi e sempre meno chiarezza. Ma c'è di più. Con questa norma sembra passare ancora l'idea dello Stato autosufficiente, smentita però dalla realtà dei fatti. Cari colleghi, il nostro Stato deve dimostrare di poter rimborsare il suo debito, come tutti, soprattutto poi se gli investitori sono in maggioranza stranieri. È proprio la relazione con i mercati internazionali che ha determinato diversi limiti alla spesa pubblica. Tali limiti - lo sappiamo - sono correlati a conseguire nel lungo periodo la sostenibilità e il rientro dal debito. Per tali ragioni, non a caso, gli Stati dell'Unione europea hanno firmato un trattato internazionale, n. 243 del 2012, che oggi ci apprestiamo a modificare. Così - come è noto - si è introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio, di cui tanto si è parlato e si continua a parlare. Cosa significa tutto questo in termini concreti? Cosa significa per i cittadini e per chi ci amministra? Significa che quei passaggi hanno prodotto notevoli restrizioni per gli enti locali anche sul piano della loro legittima autonomia. Parlare di restrizioni per Comuni, Province e Città metropolitane poi vuol sempre dire disagi e limitazioni per i cittadini. Inoltre, non è stato possibile incorporare le novità legate alla riforma della contabilità pubblica. Di certo, perciò, è opportuno modificare la legge n. 243 del 2012, superando i limiti del disegno iniziale. È opportuno per assicurare una maggiore flessibilità nella gestione dei contributi per risanamento e crescita. Allo stesso tempo, però, come dicevo all'inizio del mio intervento, l'ennesimo cambiamento del quadro normativo colpisce i nostri amministratori e la possibilità di programmare in tempo e con regole certe. Spendo allora, ancora una volta, una parola in difesa degli amministratori locali, accusati spesso in male fede di non pianificare bene le proprie «politiche». Lo faccio rivolgendomi senza mezzi termini al Governo, che è parte in causa in questa sterile polemica. Troppe volte dal Governo si è detto che la colpa dell'aumento della spesa pubblica è degli enti locali. Scusatemi, ma sono ed erano inutili *slogan* per mascherare le vere fonti dello spreco. Se questo Governo avesse voluto, avrebbe realmente cancellato le Province, ma non lo ha fatto. Smettiamola allora con la politica degli *slogan* e smettiamola di fare il tiro al bersaglio nei confronti degli enti locali. Chi maltratta gli enti locali, maltratta i propri cittadini! E chi lo fa - lo ripeto - sa fare solo propaganda, senza alcun legame con la realtà. Secondo un recente studio nazionale di pochi giorni fa, il debito degli enti locali è diminuito del 14 per cento, mentre la spesa centrale è salita del 5 I Comuni, ad esempio, negli ultimi ventiquattro mesi hanno ridotto il loro debito di ben 3 miliardi. Al contrario, il debito dello Stato è cresciuto. Per tali ragioni, ricordo a quest'Assemblea e a chi ci ascolta che ho proposto, a partire dal bilancio di esercizio del 2017, misure per rilanciare gli investimenti locali faticosamente avviati con la legge di stabilità 2016. Ho chiesto poi di redistribuire i vincoli di finanza pubblica su scala nazionale. Tutto ciò al fine di prevedere un giusto meccanismo di solidarietà nazionale e l'utilizzo *in toto* delle risorse disponibili. Capite bene che tale visione è opportuna per tenere unito ed efficiente il nostro Paese. Tale visione è inoltre strategica per consentire la tanto desiderata spinta agli investimenti locali, senza la paura degli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tale visione - e concludo, cari colleghi - è necessaria per sperare che la politica, oltre che con i numeri, sappia fare i conti con la vita e i bisogni delle persone che abitano le nostre comunità. Non dimentichiamolo!

la legge n. 243 del 2012, che effettivamente imponeva agli enti locali dei vincoli molti stringenti. Pensate che un ente locale doveva rispettare addirittura quattro

il Governo Letta, per accordi vari, è stato costretto a toglierla. Mi sembra che Renzi non fosse ancora il Presidente del Consiglio, ma era il segretario

ad andare incontro alle esigenze degli enti locali. Prendiamo ad esempio le Province: anche in questa sede abbiamo sentito spesso

anche in questo caso, ha detto: avete visto come sono bravo, ho fissato nuovi livelli essenziali di assistenza. A scapito di chi, però? Delle Regioni.

chiarito che l'intervento statale nei confronti delle autonomie territoriali non deve alterare il rapporto tra fabbisogni complessivi e insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte, né determinare squilibri squilibri economici e finanziari degli enti, cosa che invece si sta realizzando con il disegno di legge in esame, omettendo di garantire loro le risorse aggiuntive rispetto a quelle riferite per l'esercizio delle normali funzioni. Questo è un po' il voler calpestare le autonomie, gli enti locali, le Regioni, le Province

Nell'ultimo quinquennio la riduzioni di risorse e l'inasprimento dei vincoli del Patto di stabilità ha contribuito per circa 12 miliardi di euro al conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. Questo si è reso possibile perché nella finanziaria 2016 non sono stati previsti ulteriori tagli alle risorse, ma anzi sono stati concessi significativi spazi di manovra sul fronte degli investimenti, per effetto dell'abbandono del Patto di stabilità interno, sostituito dal nuovo saldo di competenza finale. per poter esplicare appieno le proprie potenzialità espansive, necessita di ulteriori interventi normativi che ne consentano il consolidamento, primo fra tutti la revisione dei vincoli di bilancio disciplinati dall'attuale formulazione della legge n. 243 del 2012. Modificare la legge n. 243, in particolare il Capo IV relativo alla finanza locale, è un canale obbligato per superare i limiti del disegno iniziale. Si sente veramente il bisogno di una sistemazione normativa che consenta di assicurare un assetto finalmente stabile della finanza comunale, da troppo tempo oggetto di numerosi interventi, che hanno compromesso la capacità programmatoria della maggior parte delle nostre amministrazioni. Gli enti locali italiani devono essere posti in condizione di operare in un contesto di regole certe e stabili nel tempo. Queste modifiche, particolarmente attese dalle Regioni e dagli enti locali, riguardano le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali, le disposizioni inerenti il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali ed infine le disposizioni relative al concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Certamente è ritenuto apprezzabile il passaggio dai quattro saldi ad un saldo unico non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto, ma non si può sottacere che il problema più importante, che preoccupa gli enti territoriali, riguarda l'eventuale utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, che la legge finanziaria 2016 (al comma 711

un emendamento che prevede una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale il fondo pluriennale è introdotto con la legge di bilancio, mentre a decorrere dal 2020 lo stesso sarà introdotto definitivamente tra le entrate e le spese finali. Molto rilevante per la gestione del debito locale è la revisione apportata all'articolo 10 dell'attuale legge n. 243 del 2012. Alla luce delle modifiche promosse dal testo, le operazioni di indebitamento non dovranno più essere soggette, infatti, alla verifica di un saldo finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione. Tale modifica favorirà certamente l'utilizzo del debito e le operazioni di investimento finanziate con gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, attraverso apposite intese da concludere in ambito regionale, che dovranno garantire in ogni caso il rispetto del saldo finale di competenza a livello aggregato. Pur apprezzando i passi avanti compiuti con questo provvedimento, che certamente segna un qualche miglioramento per la disciplina complessiva, molte altre cose andrebbero riviste e corrette, compresa la previsione di cui all'articolo 3, secondo cui lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. Ritengo che questo aspetto debba essere maggiormente rafforzato. Ancora, va ulteriormente esplicitato, migliorato e corretto l'inserimento in maniera strutturale del fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati rilevanti ai fini del nuovo saldo finale di competenza, questo sia per affrontare il tema dell'incertezza della composizione del saldo, che non darebbe stabili garanzie al rilancio degli investimenti locali, ma anche per una ragione di coerenza con la nuova contabilità. Tale criterio che rischierebbe di rimanere insoddisfatto se non si rendesse stabile e strutturata la fondamentale funzione di raccordo che il fondo pluriennale vincolato svolge tra i vari bilanci annuali, a tutto vantaggio dell'efficacia della programmazione territoriale. Inoltre, bisognerebbe affrontare in maniera più costruttiva il tema dell'*overshooting*, ovvero lo sconfinamento rispetto ad una valore che ci si è posti come obiettivo. Negli ultimi anni, infatti, gli esiti del rispetto del Patto di stabilità interno sono stati caratterizzati da margini finanziari, anche ampi, che gli enti territoriali non hanno potuto utilizzare. Quindi la portata della manovra finanziaria assegnata al comparto degli enti territoriali dovrebbe portare lo Stato a perseguire l'obiettivo di favorire, mediante specifiche misure, un pieno utilizzo della capacità di spesa consentita al sistema delle autonomie locali. Va considerato, infatti, che una quota di *overshooting* risulta fisiologica, poiché non accade mai che gli enti impegnino tutti gli stanziamenti previsti. Partendo da questo dato, quindi, è ragionevole proporre, tramite magari un'apposita norma da scrivere all'interno della legge di stabilità, la possibilità che gli enti possano utilizzare una quota parte dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese in conto capitale. Una misura di questo tipo potrebbe essere determinante per favorire certamente gli investimenti locali, senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tutto questo, unito ad una migliore redistribuzione degli spazi finanziari, potrebbe consentire davvero un sensibile passo avanti perché chi è stato amministratore di enti territoriali sa quanto sia difficile, soprattutto in tempi di crisi e assottigliamento delle risorse, scampare al rischio, terribile e sempre in agguato, del dissesto finanziario. Signor Presidente, il Gruppo che rappresento in questa dichiarazione di voto voterà in maniera diversa, a seconda delle proprie sensibilità. Per quanto mi riguarda, dichiaro il mio voto contrario.

come si dice in Toscana, cominciare dal principio, cioè con la sottoscrizione del Patto euro plus del marzo 2011, con la pistola puntata della Commissione europea e con lo spettro della *troika* che cominciava ad aleggiare. Il Patto ha inserito nel nostro ordinamento un principio per cui tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito in ossequio alle regole europee: una stretta voluta fortemente dalla Germania, e che è diventata poi il pilastro di quelle politiche di austerità declinate alla lettera in Italia dal Governo Monti e che hanno determinato le conseguenze che tutti abbiamo sotto gli occhi. Niente crescita, disoccupazione e impoverimento del ceto medio. Questo Governo si è molto impegnato in Europa, con alterne fortune, per una maggiore flessibilità di spesa nei diversi Paesi della zona euro, allo scopo di far ripartire l'economia, e ha ottenuto un primo margine di flessibilità di spesa per il 2016 per circa l'uno per cento del prodotto interno lordo: un risultato grazie al quale l'ultima legge di stabilità ha potuto abolire il Patto di stabilità interno, non prevedendo ulteriori tagli alle risorse e concedendo significativi spazi di manovra sul fronte degli investimenti. L'ANCI aveva più volte auspicato che il 2016 fosse l'anno decisivo per il superamento del Patto di stabilità, per stimolare la ripresa degli investimenti locali, sbloccando definitivamente gli avanzi di bilancio, acquisendo certezze sulla capacità di investimento ed evitando il rischio di paralisi nella realizzazione delle opere. Alcuni sindaci si erano detti pronti a violare il Patto di stabilità, nella consapevolezza che il primo volano a portata di mano per la crescita è costituito dallo sblocco del Patto di stabilità, almeno per gli investimenti e per le infrastrutture. Ad essere penalizzati erano i Comuni più virtuosi che, pur avendo soldi a disposizione, erano impossibilitati a spenderli. Molti di quei sindaci avevano non una, ma mille ragioni. Ora finalmente si supera questo paradosso, questo limite penalizzante, e l'affermazione del principio "tanto entra, tanto esce" è stato un passaggio obbligato per superare i limiti dell'interpretazione restrittiva del pareggio di bilancio in Costituzione. Questo disegno di legge, insomma, consente agli enti territoriali una gestione più efficiente delle risorse a livello locale nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, rafforza i patti regionali per incentivare maggiori investimenti sui territori. L'obiettivo di conferire un assetto finalmente stabile della finanza pubblica e di restituire un'adeguata capacità programmatoria alle amministrazioni locali va nella giusta direzione, perché gli enti locali hanno l'urgenza di poter operare in un contesto di regole certe e stabili nel tempo. La proposta del Governo ha accolto alcune modifiche attese da tempo dal sistema degli enti locali, prima fra tutte quella relativa all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243, che prevede un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali e le spese finali. Voglio rimarcare che quella sugli enti locali fu, in tutta evidenza, una parte approvata troppo in fretta nel dicembre 2012, visto che, tra le altre cose, prevedeva il rispetto da parte degli enti locali di ben otto vincoli di bilancio. Il dibattito in queste settimane si è incentrato sulla presenza - solo eventuale nel testo originario - del fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di competenza legato agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per l'anno di riferimento dalla legge di stabilità; una soluzione non sufficiente a soddisfare la necessità - peraltro più volte richiamata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge - di garantire la coerenza del vincolo finanziario con il nuovo sistema contabile degli enti territoriali. L'ANCI ha sottolineato più volte il rischio di pregiudicare la ripresa degli investimenti locali e di penalizzare proprio gli enti che hanno creduto nel definitivo superamento dei limiti irrazionali il vice ministro Morando li ha definiti "stupidi" - posti dal vecchio Patto di stabilità. Eppure, il Fondo pluriennale vincolato è stato istituito proprio per porre finalmente rimedio al problema dei residui inutilizzati dei bilanci comunali, e inserirlo o meno nel calcolo dei saldi di anno in anno con le leggi di stabilità comporterebbe grandi difficoltà proprio sugli investimenti, rendendo impossibile la programmazione delle spese con un orizzonte superiore a quello di un anno. Tutto si cambia perché nulla cambi, del resto, è una consolidata tradizione italiana, ma gli emendamenti approvati in Commissione bilancio all'unanimità hanno almeno in parte scongiurato questo rischio, rispondendo all'esigenza di una maggiore flessibilità con la previsione di una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale il fondo pluriennale vincolato sarà introdotto fra le entrate e le spese finali secondo quanto stabilito con la prossima legge triennale di bilancio. Al termine del bilancio triennale 2017-2019 si entrerà in una fase a regime in cui il fondo pluriennale vincolato sarà introdotto in via permanente fra le entrate finali e le spese finali degli enti territoriali. Una novità sicuramente positiva è rappresentata poi dal meccanismo di incentivazione per le amministrazioni locali che rispettano i vincoli di finanza pubblica: una nuova visione rispetto al recente passato, quando si prevedevano solo sanzioni. In conclusione, la normativa della contabilità pubblica deve essere stabilizzata per favorire l'efficienza e la trasparenza dei bilanci annuali, in modo da agevolare la programmazione degli enti locali e lo sblocco degli investimenti che possono contribuire in modo decisivo alla crescita dell'intero Paese. L'obiettivo di garantire un realistico equilibrio dei conti senza compromettere la capacità di spesa e di investimento dei Comuni serve a far funzionare in modo strutturale il pareggio di bilancio "semplificato" introdotto dalla manovra 2016 che ha messo in soffitta il vecchio Patto di stabilità. Dopo un ventennio caratterizzato da un contributo quasi insostenibile dei Comuni al risanamento dei conti dello Stato (13 miliardi solo negli ultimi cinque anni) e da un conseguente drastico calo degli investimenti, con la legge di stabilità 2016 e con questo disegno di legge si sono poste le basi per una ripresa effettiva, in coerenza con la maggiore flessibilità chiesta dal Governo all'Europa. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo AL-A. Presidente, la valutazione che diamo di questo provvedimento è parzialmente positiva nella parte che consente al sistema delle autonomie locali e alle Regioni di avere una maggiore possibilità di manovra finanziaria e di subire conseguenze per qualche misura ridotte rispetto grazie. Manteniamo in via generale le riserve che stanno a monte di queste misure di armonizzazione dei bilanci e di ricerca ansiosa di un equilibrio tra entrate e spese, accompagnate da una valutazione sulla sostenibilità del debito che è sempre deficitaria sotto il profilo degli effetti positivi che politiche di investimento coraggiose potrebbero determinare sull'andamento economico e quindi, conseguentemente, anche sulle entrate dello Stato. Queste riserve hanno origine all'accettazione, secondo noi passiva, di quel quadro politico molto ampio

perché quello è il peccato originario da cui discende tutta la normativa conseguentemente adottata ai fini del raggiungimento di quel riequilibrio tra entrate e spese e sostenibilità del debito, di cui abbiamo detto. Per cui un'attenuazione di quella normativa è sempre positiva. La ragione per la quale ci troviamo di fronte a questo impianto

dai primi accenni di crisi che hanno colpito il sistema economico occidentale, quello europeo e quello italiano in particolare, e il crollo della possibilità di crescita, tanti punti di PIL persi, si è accompagnato a processi di impoverimento significativi del sistema economico nazionale e economico nazionale e anche a un impoverimento complessivo della condizione di vita dei nostri cittadini e delle nostre famiglie. Non

della Costituzione e alle norme che ne sono conseguite, non ha determinato né una significativa riduzione del debito (noi abbiamo un debito in rapporto al PIL veramente esagerato), esagerato), né un'inversione di tendenza nell'andamento della crescita economica. Noi stiamo venendo da un periodo di recessione acuta, siamo in un periodo di sostanziale stagnazione, abbiamo anche preoccupazioni gravi per le condizioni in cui versa lo stato delle relazioni internazionali, abbiamo una grave preoccupazione di poter tornare in un periodo di recessione acuta. A questa partita bisogna quindi dare una risposta e il sistema pubblico nel suo complesso con l'utilizzo della finanza pubblica, anche attraverso il sistema delle Regioni e degli enti locali, locali, è strategico e va rivisto. Noi non possiamo vivere cercando di mantenere lo *status quo*. Dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza, ricostruire una prospettiva di sviluppo economico, avere un'idea del sostanziale rilancio della nostra economia e della vita, e della vita, di un nuovo sviluppo che riguarda le nostre comunità, poggiando proprio questo percorso su una nuova idea di sviluppo locale, sul radicamento di un progetto di economia che, anziché essere calata dalle centrali tecnocratiche internazionali e nazionali, è espressione di un dispiegamento di energie che parte dai luoghi, dalla necessità cioè di rispondere al raggiungimento di condizioni di vita migliori. Per fare questo, il sistema delle autonomie locali e delle Regioni è essenziale. Certo, va bene amministrato. Nessuno dice che si debba sprecare, nessuno dice

per invertire quella tendenza, per tornare a crescere, per migliorare le condizioni della finanza pubblica, per dare una prospettiva a questo Paese che non sia quella del mantenimento di un'agonia progressiva nella quale il sistema economico ma anche quello istituzionale e le condizioni sociali di questo Paese vanno verso una situazione di crisi

il sistema privato non fa investimenti, lo abbiamo detto e lo abbiamo sentito anche prima. Il sistema privato dei capitali è sempre più proiettato verso le speculazioni su se stesso (è così, è una realtà) e impoverisce tutti; quindi per muovere abbiamo bisogno di dare nuovamente capacità di intervento in economia al sistema pubblico, incominciando dagli enti locali e dalle Regioni. Questo richiama maggiore attenzione ai processi di corruzione che sono in corso anche in queste ore, ai fenomeni disgraziati con i quali siamo andati alla gestione spregiudicata della risorsa pubblica, alla mancanza di rispetto per il sacrificio di tanti lavoratori che contribuiscono a costituire quella finanza pubblica e a dare risorse. Tuttavia, fatto questo, dobbiamo rilanciare l'economia, anche utilizzando tutte le potenzialità del del nostro sistema delle autonomie locali. Se facessimo le ferrovie che devono essere fatte e spendessimo le risorse che abbiamo, se agevolassimo questo percorso,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da alcuni anni, col sopraggiungere della crisi economica, il legislatore ha posto numerosi vincoli agli enti pubblici sulle modalità con le quali utilizzare il denaro pubblico o garantire un equilibrio un equilibrio delle entrate e delle spese. Lo stratificarsi delle normative ha causato molto spesso un progressivo appesantimento del contesto operativo delle Regioni e degli enti locali, privandoli grazie. Tutto ciò ha provocato un progressivo stallo, se non un inaridimento delle politiche di sviluppo territoriali, in mancanza delle quali anche il territorio più ricco potrebbe subire perdite economiche di notevole rilevanza. Il provvedimento al nostro esame, per il quale preannuncio il voto favorevole di Area popolare, ha lo scopo di semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento raccordando le norme approvate in questi anni; semplificare le disposizioni specifiche sulla destinazione dei livelli di equilibri di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali consentendo altresì una politica espansiva; semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, dall'altro, le modalità del concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2014. Senza entrare nel dettaglio del provvedimento su cui già si è soffermata in modo esaustivo la relatrice, che ringrazio per l'egregio lavoro svolto, mi limito a sottolineare gli aspetti salienti del lavoro in Commissione e le finalità del provvedimento. Attraverso una serie di modifiche alle disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012, si vuole consentire agli enti territoriali, mediante l'attribuzione di strumenti di finanza pubblica coerenti con il nuovo ordinamento contabile, una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, tenendo conto delle specificità di ciascun ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio, sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle Regioni quale cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento. Sottolineo questo punto perché estremamente rilevante: sino ad ora non si comprendeva perché un ente virtuoso non potesse utilizzare i propri avanzi di amministrazione per politiche di sviluppo. Con questo provvedimento garantiamo questa opportunità. In tema di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, il testo originario del provvedimento disponeva, inoltre, l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica,

fondati sull'esigenza di includere tale fondo in via permanente fra le entrate e le spese finali, è stato approvato all'unanimità un emendamento della relatrice che, nel merito, prevede una fase transitoria, per gli anni 2017-2019, durante la quale il fondo pluriennale vincolato è introdotto con legge di bilancio, e la definitiva inclusione dello stesso, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali. L'utilizzo del fondo pluriennale vincolato determina una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto. Sempre per garantire maggiore elasticità agli enti locali, viene soppresso il vincolo, previsto a legislazione vigente, di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione del debito maturato dell'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci. Infine, si prevede che con legge dello Stato siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle Regioni, ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo in esame. Nella versione vigente non sono previsti premi, ma soltanto sanzioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale. In sede di esame del provvedimento in Commissione bilancio è stato approvato all'unanimità dalla Commissione un emendamento della relatrice con il quale si prevede che le operazioni di indebitamento e di investimento realizzate dagli enti locali attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base di appositi patti di solidarietà nazionale. La norma introduce un livello nazionale di rimodulazione dei saldi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, facendo ovviamente salvi gli effetti di tale strumento nazionale rispetto all'invarianza del saldo finale del complesso degli enti territoriali. Infine, il Governo ha accolto in sede di esame del provvedimento presso la Commissione bilancio un ordine del giorno che lo impegna ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che consenta ai Comuni di utilizzare l'avanzo di amministrazione per raggiungere il pareggio di bilancio, evitando il passivo e il dissesto finanziario. Auspico che a questo impegno impegno venga data un'attuazione immediata da parte del Governo. Dopo l'*austerity* più intransigente, si dà finalmente maggiore respiro ed autonomia agli enti territoriali più virtuosi. Questa è la strada da perseguire con forza e tenacia. Area Popolare la persegue convintamente, manifestando il proprio pieno assenso al provvedimento. *(Applausi

in fedele attesa da oltre due anni. Poi sono andata avanti e ho voluto contestualizzare questo provvedimento. Se è vero che gli enti locali adesso potranno utilizzare i loro avanzi per gli investimenti, bisogna vedere come vengono trattati gli enti locali. Mi sono ricordata di una tabella del DEF che abbiamo approvato qualche mese fa.

Mentre quello delle amministrazioni locali passerà da 140.000 a 126.000. Qui l'intenzione non è quella di agevolare gli investimenti, ma è la solita, ovvero quella di dare a Renzi e al Governo centrale la possibilità di usufruire della flessibilità europea, quando riesce a conquistarla, per le marchette elettorali delle prossime elezioni, per il *bonus* bebè, per il *bonus* degli 80 euro, per il *bonus* Stradivari, per i *bonus* vari a comprare voti

Prima avevamo infatti un fondo, che garantiva l'intervento dello Stato, ma adesso, come è prassi del Governo Renzi, si delega ad altre leggi ordinarie, che è come dire che non si farà nulla. Questo vuol dire ciò. Il principio della delega ormai governa il nostro Paese, quando vuole e può, magari di notte, come ha fatto con Banca Etruria, di domenica sera e di nascosto, allora il Governo emana i provvedimenti, che altrimenti rimangono chiusi in un cassetto.

meno: è un po' come facciamo noi in Europa, quando andiamo lì a mendicare. Siccome l'Europa ormai è diventata altamente politica, perché si occupa solo di salvaguardare il proprio potere, essa dà la possibilità di produrre nuovo debito pubblico, che poi ci teniamo sul groppone

Quindi, dopo aver contestualizzato questo ennesimo *spot* del Governo Renzi, il Movimento 5 Stelle decide convintamente di votare «no» al provvedimento in esame, perché siamo contro il *fiscal compact*, siamo contro le regole europee, siamo contro un' Europa che è fuori dal controllo dei cittadini, siamo contro un Governo prono, che accetta pedissequamente di fare ciò che l'Unione europea ci impone. Noi vorremmo invece allentare veramente le maglie e se c'è da fare debito pubblico, che si faccia, che si aggiustino le scuole, che si investa nella tecnologia, nella ricerca, nell'università, nella lotta al dissesto idrogeologico, che si investa nei trasporti e che non si piagnucoli dopo, con le facce da circostanza, in televisione, perché infame e indecente! Almeno abbiate la decenza del silenzio, perché avete piene responsabilità su quello che succede. Non demandate all'errore umano! Qui non c'è nessun errore umano.

Questa è la verità. Alzate la testa, anche voi, amici della Lega, e aprite gli occhi, perché è una dinamica che vuole che il Sud rimanga povero. Questa è la verità. verità. Il Movimento 5 Stelle, anche questa volta, e per l'ennesima volta, dichiara un voto contrario per questioni non soltanto di principio, ma anche di merito. Ricordatevelo quando ci saranno gli effetti di questo disegno di legge, perché siete stati voi, uno alla volta, a votare di nuovo il *fiscal compact* compact* per gli enti locali. Non vi meravigliate o non date retta a Renzi che dice che i Governi precedenti avrebbero dovuto salvare le banche e non avrebbero dovuto adottare il *fiscal compact*. Siete voi, qui, che lo state votando ancora e ancora. Con spirito di collaborazione, abbiamo presentato numerosi emendamenti, proponendo le modifiche che ritenevamo necessarie e che abbiamo individuato attraverso un confronto a tutto campo con gli amministratori locali. L'atteggiamento del Governo e del partito di maggioranza è stato, però, chiaro e netto: non ci serve nulla, nessun parere favorevole, nessun nostro emendamento approvato. signor Ministro, il dialogo con gli enti locali è fondamentale per la tenuta delle istituzioni. Gli enti locali sono il *front office* delle istituzioni e non potete continuare a trascurare le loro esigenze e richieste. Gli enti locali stanno sopportando e sostenendo un grande sforzo per far fronte alla grave crisi economica che sta strangolando il Paese e che voi continuate a negare. Gli enti locali hanno il problema non solo delle regole per utilizzare le risorse, ma anche della quantità delle risorse disponibili che continuano a diminuire. ultimi anni il Governo - proprio questo Governo che ha come *Premier* un ex sindaco e che ai sindaci ha fatto sempre riferimento come modello a cui ispirarsi - ha ridotto drammaticamente i trasferimenti ai Comuni italiani. I Comuni hanno reagito con responsabilità e serietà, diminuendo nel solo biennio compreso tra l'aprile del 2014 e il marzo del 2016 i propri debiti di ben 3 miliardi di euro. Peccato che, nel frattempo, il debito dello Stato centrale sia aumentato di ben 96 miliardi E oltre al danno la beffa, perché avete obbligato i sindaci ad aumentare le tasse locali per poter sopravvivere, scaricando su di loro una responsabilità che - invece - è solo vostra e l'avete fatto solo per poter dire che avete abbassato le tasse, ben sapendo che questa è l'ennesima bugia.

Contemporaneamente, la crisi ha determinato un forte aumento delle richieste dei cittadini che si rivolgono ai Comuni per superare le loro difficoltà. Chi è in difficoltà, e non riesce a pagare la bolletta dell'acqua, della luce e del gas e non ha risorse per mangiare o addirittura per curarsi, si rivolge al Comune. Sono i Comuni - ad esempio - che assistono e sostengono i costi per i minori che entrano in Italia attraverso un'immigrazione scriteriata e inarrestabile e che vengono affidati alle strutture di accoglienza. Nel 2015 si è trattato Il Governo deve ascoltare con più attenzione il grido di allarme sulla condizione e le problematiche quotidiane che vivono gli enti locali. Voi state troppo nel Palazzo, viaggiate con l'auto blu e la scorta e non vi rendete conto della drammatica situazione in cui vive il Paese. Non vedete in che condizione di incuria sono ridotte le strade provinciali e comunali, nelle quali non si sfalcia più l'erba sulle scarpate e non si effettua più la potatura degli alberi. Quando piove, le strade sembrano torrenti, con l'acqua che attraversa e invade la carreggiata, con rami che cadono sulle auto in transito, determinando gravi pericoli per gli automobilisti e a volte incidenti anche mortali. Gli asfalti sono pieni di buche, tanto da renderli pericolosi al transito. Sarà per puro caso che sono tornati ad aumentare gli incidenti stradali o ci sono delle vostre responsabilità? Questo provvedimento di legge di iniziativa governativa del ministro dell'economia e delle finanze Padoan contiene modifiche all'ordinamento finanziario degli enti locali che non risolvono alcun problema. La necessità di consentire agli enti territoriali di gestire le risorse in modo più efficace, tenendo sempre conto delle singole specificità e rispettando gli equilibri di bilancio, nonché di favorire gli investimenti sul territorio, potendo ricorrere al debito oppure mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, non è affatto soddisfatta. il consolidamento del ruolo delle Regioni, in qualità di cabina di regia sul territorio, è un ostacolo all'autonomia dei Comuni. Ma vi pare utile o opportuno e ragionevole che, per utilizzare un avanzo di amministrazione, cioè soldi propri degli enti locali, un ente debba acquisire un'intesa regionale? Rimangono ancora in piedi parecchie perplessità in merito all'esercizio in corso, ed eventualmente anche a quelli futuri, cui la modifica della legge n. 243 del 2012 doveva dare consistenti e durevoli risposte che invece non dà. Ad esempio, che senso ha rinviare a un prossimo provvedimento la possibilità di consentire ai Comuni di utilizzare l'avanzo di amministrazione per raggiungere il pareggio di bilancio, evitando il passivo dissesto finanziario? Che cosa contano gli ordini del giorno? Il Parlamento è lastricato di ordini del giorno che non producono alcun effetto. Ve lo ha detto chiaramente anche il presidente dell'ANCI Fassino, che, in una lettera al ministro Padoan, ha sostenuto la necessità inderogabile che il fondo pluriennale vincolato sia inserito stabilmente e non deciso anno per anno a ogni legge di stabilità. Perché avete mantenuto questa scelta di incertezza e di provvisorietà, che impedisce ai Comuni di affrontare seriamente il problema degli investimenti e delle spese pluriennali? Avremo a breve l'ennesima modifica, sicuramente la recepirete la prossima volta. Ma voi pensate che con le leggi si possa giocare? Non oso immaginare quello che fareste con una sola lettura, così come avete previsto nella vostra riforma costituzionale. Sono convinto che questo provvedimento risolva poco e non migliori le condizioni degli enti locali, che hanno bisogno di ben altro. Gli enti locali hanno bisogno di meno regole, di semplificazioni. Di regole oramai oramai ne abbiamo troppe e nessuno le rispetta più; solo i fessi rispettano le regole. Avete eliminato le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità a Città metropolitane e Province (con l'articolo 7 del 2016, n. 113), ma avete ridicolizzato i Comuni, che hanno fatto salti mortali per rispettare il Patto nell'anno passato. Possono continuare gli enti locali a pagare tassi di interesse sui mutui con le banche o con la Cassa depositi e prestiti del 5-6 per cento (tassi di usura), quando i tassi correnti sono addirittura sotto zero? Ma vi chiedete come mai gli investimenti lordi dei Comuni sono diminuiti di più del 25 per cento negli ultimi quattro anni e continuano ancora a diminuire? I mutui contratti dagli enti locali e gli investimenti non servono per andare in vacanza, ma sono gli strumenti che i Comuni utilizzano per realizzare strutture e servizi per il cittadino. Per concludere, siamo di fronte a un provvedimento minimo, niente di più di una pezza, utile a rimediare ad alcuni errori della legge precedente, ma che non ha l'ambizione che invece sarebbe stata necessaria per riscrivere globalmente le regole complessive dei bilanci regionali e degli enti locali, semplificando e agevolando, ad esempio differenziando tra enti di dimensione diversa. Non è possibile che per il Comune di Bolognola, che ha 150 abitanti, debbono valere le stesse regole del Comune di Roma, che ha 3 milioni di abitanti. Rimane l'amarezza che si poteva fare di più, molto di più e meglio, se solo il Governo e il Partito Democratico avessero accettato di confrontarsi seriamente con le opposizioni nel merito del provvedimento. Per le ragioni esposte, esprimiamo un giudizio critico sul provvedimento. Solo per grande senso di responsabilità il nostro voto sarà di astensione, sperando che il Governo voglia affrontare in maniera concreta i problemi degli enti locali non attraverso nuove e ulteriori regole, ma con le risorse necessarie per evitare un tracollo tracollo economico che oramai diventa irrecuperabile.

supera definitivamente il meccanismo del Patto di stabilità interno e libera, seppure progressivamente, maggiori spazi finanziari per le amministrazioni locali. Le misure al nostro esame si inseriscono in un percorso già avviato con la legge di stabilità 2016, provvedimento con il quale è stato posto termine a una lunga fase di restrizione finanziaria operata nei confronti del comparto degli enti territoriali. Tra riduzioni di risorse e inasprimento dei vincoli del Patto di stabilità, resi ancora più ardui in ragione della crisi economica, gli enti territoriali nel corso dell'ultimo quinquennio hanno dato un decisivo contribuito al conseguimento dei difficili obiettivi di risanamento della finanza pubblica. La legge di stabilità 2016, per la prima volta dopo molti anni, non ha previsto ulteriori tagli alle risorse degli enti locali ma, al contrario, ha concesso significativi spazi di manovra sul fronte degli investimenti. Con la manovra 2016 è stato riconosciuto agli enti territoriali un nuovo ruolo istituzionale, fondamentale per agganciare la ripresa economica. - questo è il punto di oggi - l'impianto della legge di stabilità 2016, per poter esplicare appieno le proprie potenzialità, necessita di ulteriori interventi normativi che ne consentano il consolidamento, a cominciare dalla revisione dei vincoli di bilancio disciplinati dall'attuale formulazione della legge n. 243 del 2012, che sono appunto l'oggetto del nostro provvedimento. La legge n. 243 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento, in modo costituzionalmente rafforzato, obblighi di pareggio di bilancio derivanti dalla situazione di gravissima instabilità della finanza pubblica che il Paese ha affrontato dalla fine del 2011. L'impostazione della legge n. 243, fondata sull'imposizione di obblighi e vincoli da applicare indistintamente a ogni singolo ente locale, ha delineato un assetto finanziario degli enti territoriali rigidamente regolato. Ora, superata la fase di crisi acuta della finanza pubblica, le modifiche introdotte alla legge n. 243 superano diverse rigidità e difficoltà applicative del testo attualmente vigente. Esse mirano a una profonda revisione degli obblighi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, con l'esplicito obiettivo di pervenire a un quadro di vincoli coerenti rispetto alle nuove regole della contabilità pubblica. La modifica di più consistente interesse per gli enti territoriali è, senza dubbio, quella relativa al comma 1 dell'articolo 9. In linea con quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, la nuova disposizione sostituisce i quattro vincoli di competenza

a partire dal 2020, tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di competenza. E questo è un passo avanti molto importante, e ringrazio nuovamente tutti i Gruppi che hanno sostenuto la nostra proposta. Da questo punto di vista siamo a un passo importante anche rispetto alle aspettative dell'Unione dei Comuni e degli altri enti territoriali. È questa una soluzione che soddisfa la necessità di garantire la coerenza del vincolo finanziario con il nuovo sistema contabile e la formulazione è destinata a favorire una decisa ripresa degli investimenti locali, che ha tra i suoi presupposti proprio l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel nuovo saldo recata dalla legge di stabilità. La stabilizzazione di questa declinazione del saldo di competenza, nel quale viene incluso anche il fondo pluriennale vincolato, è un obiettivo essenziale

il Partito Democratico ritiene molto importante che la prossima legge di bilancio faccia lo forzo massimo affinché il fondo pluriennale vincolato venga inserito in misura molto consistente, e nell'arco del triennio in modo completo, nel saldo tra entrate e uscite, così da dare a questa norma la forza che essa deve sviluppare per favorire la ripresa del Paese e degli investimenti. Molto rilevante per la gestione del debito locale è anche la revisione apportata all'articolo 10, che favorirà l'utilizzo del debito e le operazioni di investimento finanziate con gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, attraverso apposite intese da concludere in ambito regionale. Qualora tali operazioni non siano soddisfatte dalle intese regionali, le stesse sono effettuate sulla base di appositi patti di solidarietà nazionali, introducendo di fatto un livello nazionale di rimodulazione dei saldi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali. Nel complesso, le modifiche consentiranno di semplificare notevolmente le procedure di ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento degli enti territoriali e la realizzazione di interventi nel territorio. Altre importanti modifiche si riferiscono alle azioni che lo Stato potrà attuare nei confronti delle autonomie territoriali in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. In conclusione, il provvedimento che ci accingiamo a votare deve essere considerato come parte fondamentale di una più ampia sistemazione normativa per assicurare un assetto finalmente stabile della finanza degli enti territoriali. Le amministrazioni locali, con l'approvazione del provvedimento, sono poste in condizione di operare in un contesto di regole certe e stabili nel tempo, restituendo a questo importante comparto una situazione di "normalità" gestionale e, soprattutto, di organizzazione e programmazione certa delle misure e degli interventi da adottare per il loro territorio. A queste, nei prossimi mesi e anni, andranno aggiunti altri robusti interventi, soprattutto in materia di semplificazioni e di decisioni ordinamentali. sottolineando il proficuo lavoro svolto durante l'*iter* del provvedimento al Senato che ha visto il contributo di tutti, maggioranza e opposizione, in un clima di collaborazione -

le soluzioni migliorative che qui oggi possiamo portare anche con una certa convinzione e con molta consapevolezza. Per tali ragioni, mi rivolgo alle senatrici

La facoltà riconosciuta al prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento, si configura certamente come diritto potestativo e in forza di tale previsione la Presidenza non ha alcun potere specifico né rispetto ai senatori, né rispetto all'Assemblea, né rispetto alla Conferenza dei Capigruppo. La prassi parlamentare ha senz'altro confermato tale interpretazione, arricchendola tuttavia di ulteriori specificazioni, sia in senso restrittivo, sia in senso estensivo. Tra queste ultime rientra la casistica per la quale, anche in assenza del prescritto numero di otto senatori, la Conferenza dei Capigruppo possa comunque provvedere all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno. Tra le specificazioni di segno restrittivo rientrano invece due distinte tipologie. La prima: laddove il Governo intervenga nell'ambito dell'oggetto trattato in seduta, ancorché al di fuori della ordinaria e prevista cadenza che il Regolamento riserva ai rappresentanti dell'Esecutivo, non si integrano i presupposti materiali della fattispecie di cui all'articolo 105 del Regolamento. La seconda: quando il Governo non interviene in via primaria, ma esclusivamente in risposta a sollecitazioni formulate da senatori, non ampliando lo spettro contenutistico degli interventi che l'hanno preceduto, la partecipazione al dibattito del rappresentante dell'Esecutivo non si qualifica come "comunicazioni del Governo" in senso proprio. Alla luce di tali considerazioni, la Presidenza rileva che l'intervento del senatore Pizzetti è stato successivo a quello dei senatori che hanno sollevato la questione principale, la quale non era di per se stessa originariamente iscritta all'ordine del giorno. Le osservazioni del rappresentante del Governo sono riconducibili a mera risposta data dall'Esecutivo alle richieste dei senatori, corredata da valutazioni che appaiono speculari ai rilievi critici sviluppati nel corso degli interventi che l'hanno preceduta. Rispetto ai presupposti di fatto della fattispecie disciplinata dall'articolo 105 del Regolamento, secondo la prassi interpretativa dianzi richiamata, difetta l'elemento cosiddetto oggettivo

se il sottosegretario Pizzetti si fosse limitato a rispondere alla questione posta dalla senatrice Bonfrisco e a seguire da una serie di altri senatori. Nel momento in cui, invece, il sottosegretario Pizzetti parla di Costituzione,

perché è evidente che comunque il sottosegretario Pizzetti non è intervenuto in fase di replica né per esprimere un parere.

Poiché l'informativa del Governo sul disastro ferroviario avvenuto in Puglia è prevista per le ore 18,30, sospendo la seduta.

Ieri, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, nel giorno del dolore e delle lacrime, durante la visita ha detto che questi sono i momenti della vicinanza alle famiglie, ma ha anche aggiunto che è necessario fare chiarezza al più presto. Su questo garantiamo garantiamo tutta la nostra collaborazione e il nostro impegno per coadiuvare i magistrati inquirenti e la Regione Puglia, che non lasceremo sola. Non lasceremo soli i suoi sindaci, cui continueremo, anche nelle prossime settimane, a stare accanto. L'incidente è avvenuto sulla ferrovia Bari-Barletta. È una linea ferroviaria regionale lunga 70 chilometri che collega Bari con numerosi centri abitati dislocati su due Province, che ha capolinea a Barletta e un bacino di utenza di circa 700.000 abitanti. La gestione della linea è curata dalla società Ferrotramviaria, che vi opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia d'impresa ferroviaria e che effettua anche il servizio automobilistico nel medesimo bacino. La proprietà dell'infrastruttura è della Regione Puglia. Fa parte di quel sistema di ferrovie *ex* concesse andate in gestione alle Regioni. La linea è elettrificata, a scartamento normale. È a doppio binario nel tratto tra Fesca San Girolamo e Ruvo (circa 33 chilometri), mentre per i restanti 37 chilometri è a binario unico. La circolazione dei treni avviene con blocco automatico bidirezionale da Bari a Ruvo mediante l'apparato centrale elettrico a itinerari (ACEI) e gli apparati centrali statici (ACS) di Terlizzi e Ruvo, e con blocco telefonico da Ruvo a Barletta. Il giorno 12 luglio, alle ore 11,38, si è verificato uno scontro frontale tra due convogli ferroviari della lunghezza di circa 80 metri. I convogli erano di recente produzione e immissione in servizio sulla tratta a binario unico Corato-Andria di questa linea ferroviaria gestita dalla società Ferrotramviaria. Il bilancio

La società Ferrotramviaria ha ovviamente interrotto la circolazione nella tratta. A seguito dell'incidente frontale occorso, il Dipartimento della protezione civile, avendo appreso alle ore 11,42 della notizia dell'incidente pervenuta alla Sala Situazione Italia della struttura operativa dei Vigili del fuoco, si è attivato immediatamente per seguire e valutare la portata dell'incidente, per verificare che tutto il sistema nazionale di Protezione civile fosse informato e portare da subito supporto alle autorità locali e alla Protezione civile regionale. Successivamente, sulla base delle informazioni assunte e nel rispetto delle indicazioni della normativa di settore, ha assunto la configurazione S2 (presidio operativo) ed è rimasto in video collegamento costante con il centro operativo dei Vigili del fuoco del Viminale e, attraverso la Sala Situazione Italia, con tutte le sale operative nazionali, nonché con la Regione Puglia e le due prefetture interessate. Date le rilevanti proporzioni dell'incidente, nella giornata di ieri sono state avviate alle cure ospedaliere 52 persone, di cui 11 in gravi condizioni. Come ho già detto, i medici legali hanno potuto concludere solo da poco le attività di riconoscimento delle vittime: per tutta la notte si è lavorato per ricomporre le salme e, come potete immaginare, la ricostruzione delle identità è stata molto complessa. A livello territoriale, il coordinamento delle operazioni di soccorso sul posto, in raccordo con la Regione, è stato assicurato dal centro coordinamento dei soccorsi presso la prefettura di Barletta e Andria, che è stato immediatamente approntato; nei Comuni di Corato ed Andria sono stati attivati i centri operativi comunali. Al fine di fornire supporto alle attività di soccorso, la Regione Puglia, in accordo con le ASL, ha immediatamente attivato un numero per le persone che richiedono informazioni sui passeggeri. A livello A livello centrale, valutata la gravità della situazione, alle ore 15,30 mi sono recato sul posto con il capo del Dipartimento di protezione civile, un gruppo di suoi collaboratori e il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sul posto erano già presenti il presidente Emiliano, il Vice Presidente della Regione, il direttore della Protezione civile regionale, i sindaci dei territori. Successivamente, il Presidente del Consiglio, nella serata di ieri, ha raggiunto la Puglia e, dopo aver effettuato un sopralluogo sul luogo del sinistro,

sono prolungate per l'intera notte, soprattutto l'attività di rimozione dei detriti. Al fine di verificare la possibilità di accelerare la movimentazione delle carrozze, sono state impegnate sul posto le gru più adatte alle operazioni in corso ed è arrivato, nel corso della notte, un locomotore inviato dalle Ferrovie dello Stato per garantire la massima assistenza. Le attività di ricerca, inoltre, hanno permesso di recuperare la scatola nera di uno dei due treni.

soccorsi non sono stati solo tempestivi, ma anche generosissimi. Abbiamo visto una generosità straordinaria anche da parte dei cittadini pugliesi, nel momento in cui c'è stato bisogno di donare il sangue. A loro va tutta la nostra riconoscenza e il nostro

Vorrei ora informare sul tema della sicurezza. La sicurezza della circolazione ferroviaria in tale tratta è regolata tramite il meccanismo del consenso telefonico: nel regime del blocco telefonico il capostazione non può inviare un treno alla stazione successiva se non ha domandato e ottenuto dal capostazione della predetta il consenso ad inviare quel determinato treno. Quindi la sezione di linea è dunque normalmente bloccata e viene liberata per la circolazione di volta in volta, mediante il consenso all'inoltro del treno. Quindi, con tale procedura, sulla sezione di linea può essere presente un solo treno per volta. Il sistema di segnalamento con consenso telefonico, pur essendo sicuro, è certamente un sistema tra i meno evoluti. Sui 20.000 chilometri della rete ferroviaria nazionale, di cui 16.000 di competenza statale e 3.000 di ferrovie ex concesse, solo 600 sono regolati con tale meccanismo. tutta la rete di competenza nazionale è regolata con meccanismi diversi da questo. Il sistema è sicuro, ma si affida interamente all'uomo e quindi non riesce ad avere un meccanismo di "servosterzo" rispetto all'errore dell'uomo: questo è il vero limite. Le tecnologie oggi disponibili sono ovviamente molto più avanzate, ma va detto che sulla tratta a binario semplice in esame, il sistema di consenso telefonico è in uso da oltre e l'attuale frequenza dei convogli è praticamente inalterata da circa dieci anni, durante i quali non si sono evidenziati inconvenienti nell'applicazione del sistema. Il sistema - lo ripeto - è di completa responsabilità della società di gestione, Molte delle reti secondarie sono caratterizzate anche da *standard* tecnologici più evoluti: come detto, solo 600 chilometri circa adottano questo meccanismo. nella rete delle ferrovie secondarie sono ancora presenti 2.700 chilometri di linea a binario unico. Il binario unico però - lo vorrei dire con molta chiarezza ed è opinione diffusa tra tutti gli esperti - non è sinonimo di insicurezza. di rete nazionale, 9.000 sono a binario unico e sono assolutamente attrezzati tecnologicamente e mantengono un livello di sicurezza tra i più elevati nel mondo. Le ferrovie di Stato italiane hanno infatti livelli di sicurezza tra i più elevati del mondo.

Nella fattispecie, la società Ferrotramviaria è, dalla sua costituzione, una delle aziende migliori del panorama italiano in termini di efficienza ed efficacia del servizio offerto e del livello professionale degli addetti e degli interventi di ammodernamento e miglioramento dell'esercizio. La Regione Puglia, che ha responsabilità di queste tratte regionali, ha investito parecchio nell'ammodernamento tecnologico e quella in esame non era considerata tra le linee più a rischio o più devastate nel panorama, molto complesso e poco

anche i sistemi automatizzati possono essere disattivati dall'operatore, tant'è vero che l'incidente molto grave occorso in Germania fu provocato dalla disattivazione del sistema da parte di un capostazione che voleva in questo modo accelerare la circolazione ferroviaria. Quindi, i sistemi tecnologicamente più avanzanti possono essere disattivati l'errore umano è possibile anche in questo senso. Tutto questo, ovviamente, non intende anticipare alcuna delle conclusioni che la magistratura trarrà con la sua inchiesta. inchiesta. Per accertare esattamente la dinamica dei fatti e le problematiche legate alla sicurezza abbiamo subito nominato una commissione di inchiesta, che ha lo scopo di accertare le cause dell'incidente e le responsabilità nel settore della sicurezza

ai fini della sicurezza degli impianti e le verifiche e le prove funzionali per l'apertura dell'esercizio. La gestione delle infrastrutture e dell'esercizio sulla stessa rete è in capo alle società esercenti.

La figura del responsabile è rappresentata dal direttore di esercizio, il quale rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle Regioni (in questo caso è la Regione concedente) e degli enti locali e territoriali. Il direttore di esercizio risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. Il Ministero, esercitando la vigilanza sugli aspetti riguardanti la sicurezza, ha mantenuto un'interlocuzione sia con controlli regolari sull'infrastruttura, attraverso l'ufficio sia con il responsabile della sicurezza e devo dire che non abbiamo mai dovuto annotare carenze di sorta. Quindi, il gestore, gli operatori e i responsabili si sono sempre comportati in maniera adeguata agli *standard*. Certamente questo evento pone il problema, che abbiamo sollevato non oggi o negli ultimi giorni ma da sempre, di un potenziamento e di una migliore efficienza, efficacia e messa in sicurezza del sistema di trasporto pubblico italiano.

vostra attenzione. Arriviamo quindi quasi a 18 miliardi, di cui oltre 4 miliardi nel primo aggiornamento, ma altrettanti o poco di meno nel secondo, sono destinati, in maniera finalmente decisa, anche ad interventi sulle reti regionali

lo stanziamento effettivo che il Parlamento ha approvato è appunto di 9 miliardi nel 2015 e di 9 miliardi nel 2016 complessivamente. In stabilità sono stati elencati semplicemente gli stralci i lotti costruttivi che era necessario provare ad anticipare sulle linee ad alta velocità, ma quelli non rappresentano in alcun modo gli investimenti ferroviari. Torno a parlare di "cura del ferro" e ricordo che la collaborazione che abbiamo avuto in questo anno con le Regioni è stata molto intensa, proprio per colmare questo *gap* nel trasporto pubblico locale, sebbene non sia di nostra competenza diretta perché teoricamente lo Stato potrebbe fermarsi al tema del del fondo unico per il trasporto pubblico locale. Questa interlocuzione e la sensibilità di recuperare il ritardo in questo settore hanno consentito di stanziare ben 18 miliardi, di cui una parte consistente sulle linee regionali e sul potenziamento ulteriormente del trasporto cargo. Perché? Perché sappiamo che il trasporto pubblico regionale è stato la Cenerentola di questi anni e sappiamo che abbiamo cinque milioni di persone che ogni giorno, tra metropolitane e reti regionali, salgono su questi mezzi. Per questo voi, onorevoli senatori, avete approvato, insieme alla legge di stabilità, anche un programma di investimento per il rinnovo del parco mezzi rotabile, con oltre un miliardo di euro, che permetterà di sostituire la gran parte dei treni regionali vetusti. In questo caso i treni regionali erano nuovi nuovi e non è vero che erano treni non adeguati; certamente non era adeguata la dotazione tecnologica dell'infrastruttura, che consente il dialogo tra l'infrastruttura e il treno.

di nuovo di classificare alcune reti regionali come reti che devono immediatamente avere un *upgrading* in termini di sicurezza e passare dalla vigilanza dell'USTIF alla vigilanza dell'Agenzia nazionale

di questa disgrazia, ma è scaturito dalla consapevolezza che nell'ottica di un federalismo un po' più maturo, lo Stato non deve semplicemente dire «questa non è mia competenza», ma deve essere pronto a collaborare ed essere al fianco delle Regioni e degli enti locali nella promozione del trasporto pubblico locale. In conclusione, in questo giorno di dolore e di lutto così difficile, noi non abbiamo intenzione di scaricare le responsabilità su altri, né di additare i ritardi in qualche atto amministrativo o nella spesa di qualche fondo. Questo non credo che sia il momento. Il modo migliore per onorare le vittime, i familiari e il loro dolore credo sia quello di esprimere oggi, a nome del Governo, tutta la volontà

Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, questo per me non sarà un intervento come gli altri, non può esserlo. In queste ore, la mia città, Corato, insieme a quelle di Andria, Ruvo di Puglia e Barletta, insieme alla Puglia intera, stanno vivendo un momento drammatico. Cordoglio, solidarietà, generosità, operosità: sono le parole che stanno facendo il giro del mondo e che meglio descrivono l'immagine della mia terra. Dunque, qui, oggi, voglio parlare innanzitutto da cittadino, e parlerò con il dolore e la rabbia. Ventitré vite spezzate, ventitré storie, volti, nomi di uomini, donne, bambini e giovani. Non nascondo la difficoltà, signor Ministro, onorevoli colleghi, a parlarne. Provo difficoltà soprattutto perché chi, come me, ieri ha trascorso la giornata sul luogo dell'incidente, non può e forse mai più potrà togliersi dalla mente quello che ha visto. Sono immagini che nessun messaggio di cordoglio né alcun risarcimento potrà mai cancellare. Per questo motivo, è giusto chiedere innanzitutto rispetto per le vittime e i loro familiari. Una riflessione è necessaria, molto più di qualunque retorica, per tentare di non rendere vana questa immane tragedia. I miei concittadini, tutto il popolo pugliese si sta chiedendo se tutto ciò si poteva evitare. Leggo e sento che in queste ore si susseguono tante ricostruzioni, più o meno fondate, più o meno lecite; spiace che alcune di queste, oltre che non rispettare il dolore, dipingano situazioni lontanissime dalla realtà. Lasciamo le analisi alle autorità competenti, in cui riponiamo massima fiducia, perché in tempi brevi sia fatta chiarezza su quello che è accaduto: uno dei più gravi disastri ferroviari degli ultimi anni. Vogliamo che sia fatta luce; lo dobbiamo alle famiglie delle vittime, agli amici, ai conoscenti di quelle persone che ieri, tra le macerie, hanno perso la vita. Ci sarebbe tanto altro ancora da dire, forse troppo. Mi limito a dire che quel disastro è la più drammatica evidenza di un sistema che non funziona. Ma chi crede che il Sud si arrenda o possa piegarsi dinanzi a simili tragedie, sbaglia ancora una volta. Non ci arrendiamo all'orrore e al dolore; il popolo pugliese ha saputo dare prova di immensa e straordinaria generosità, solidarietà, operosità e capacità di far fronte a una lacerante ferita. Ringrazio con il cuore in mano, in quest'Aula, le Forze dell'ordine, tutte le istituzioni, i medici, la Protezione civile e i tanti volontari che da tutte le zone della Puglia sono intervenuti in soccorso della tragedia di ieri. Credo che il miglior modo per riscattare la gente scomparsa ieri sia lottare per la verità. Credo che l'unico modo utile che abbiamo per onorare quelle vittime sia proporre soluzioni concrete. Il ministro Delrio, in rappresentanza del Governo, ci dia un doveroso chiarimento. Non spetta a me, e certamente a nessuno di noi in quest'Aula oggi, attribuire delle colpe. Che si sia trattato di un errore umano o di carenze tecniche e di sicurezza è una questione sulla quale le indagini da parte della magistratura e delle autorità competenti devono fare il loro corso. Quello però che mi preme dire in quest'Aula e in particolare proprio a lei, signor Ministro, che oggi nel suo discorso alla Camera e poi anche qui ha annunciato con vivo entusiasmo lo stanziamento di ulteriori risorse a favore del trasporto ferroviario, di cui prendiamo atto, è che immettere liquidità nelle casse degli enti locali non può essere considerata la panacea a tutti i mali. Il problema non sono le risorse disponibili ma il modo in cui queste vengono adoperate o, troppo spesso, non adoperate a causa di vincoli burocratici e ostacoli legati alla finanza pubblica. Si parla da cinquant'anni di Sud e di problemi del Sud, eppure il Paese continua a correre a velocità separate. Si cominci allora dalla più urgente delle necessità: leggi chiare, norme che non diano adito a interpretazioni equivoche e a una matassa ingarbugliata di provvedimenti confusi, che rendono ancora più complessa la già faticosa vita delle amministrazioni locali. Il dramma dell'incidente ferroviario in Puglia è la più drammatica evidenza dei danni enormi che può produrre una nefasta e farraginosa macchina statale, al prezzo di vite umane. Nel 2011, da sindaco di Corato, la mia amministrazione ha approvato il progetto che prevedeva il potenziamento della rete delle Ferrovie del Nord Barese, proprio sulla tratta Corato-Barletta, che avrebbe dovuto essere ultimato utilizzando i fondi strutturali della Comunità europea della programmazione 2007-2013. Sono passati cinque anni e ancora si parla di aggiudicazione della gara d'appalto. Al di là di ogni sterile polemica e qualunque siano le responsabilità che andranno accertate in maniera celere, ciò evidenzia un imperdonabile ritardo

Di fronte a una tragedia così immane, la politica si interroghi in coscienza, a tutti i livelli istituzionali, se ha fatto la sua parte. Concludendo, e stringendomi ancora una volta alla mia Regione, chiedo a lei, signor Ministro, di trovare le parole e forse anche le ragioni per dare la più difficile delle risposte alla più banale delle domande: perché ancora accadono queste cose? Per il rispetto della Puglia, del mio popolo, e di tutti coloro che purtroppo ancora muoiono in tragedie come questa, ci dica il Governo chiaramente cosa intende fare nell'immediato.

questi eventi, che si possono definire assurdi, inconcepibili e sicuramente incomprensibili in particolare per i nostri cittadini. Ce lo siamo detti molte volte in Commissione, signor Ministro:

ai primi posti all'interno dello scenario europeo come efficienza e come rete e questo è sicuramente un fiore all'occhiello del nostro Paese, ma lei sa benissimo che quando invece andiamo a parlare di trasporto locale, purtroppo siamo agli ultimi posti e questa è un'anomalia che solo nel nostro Paese si riscontra.

Lei ha parlato della sua "cura del ferro", della quale in altre occasioni (non lo farò questa sera) ho avuto modo di disquisire per i tempi, i modi e il sistema di finanziamento.

c'è un opera, che è il raddoppio della tratta Cefalù-Castelbuono, per cui sono a disposizione più di 335 milioni di euro e i lavori non partono per

se mai ritorneremo a parlare di privatizzazione delle ferrovie. Non siamo restii a parlare di privatizzazione delle ferrovie, ma siamo

- ho già detto una volta che facciamo il tifo per lei da questo punto di vista e non per il Ministro dell'economia - sia l'occasione per rilanciare il settore ferroviario per il trasporto pubblico locale. Per il resto, signor Ministro, confidiamo di non doverci ritrovare ancora una volta

Con la stessa chiarezza le dico che invece alcuni punti del suo intervento non mi hanno convinto. Non mi convince il fatto che, poiché da il sistema dell'avvertimento attraverso telefono ha funzionato, questo non sia un elemento critico da segnalare come un inaccettabile ritardo. Vede, signor Ministro, nella mia Regione, a pochi chilometri dal dal luogo dove è avvenuto quel disastro, c'è una impresa, la MERMEC (che credo il Presidente del Consiglio conosca bene e abbia anche visitato), che è la più importante al mondo nell'ambito della sicurezza ferroviaria. Quando la si visita si rimane sbalorditi e ci si chiede come sia possibile che da un piccolo centro del Sud d'Italia si possa controllare lo

non ci può far stare tranquilli, né possiamo semplicemente limitarci a registrare il fatto che per sessant'anni sia andata bene. Questi sono ritardi dei quali dovremmo farci carico, dei quali il Governo dovrebbe farsi carico. modo lei ha assolutamente ragione nel dire che il binario unico non implica di per sé insicurezza, implica mancanza di sviluppo e di investimenti e a me non ha mai convinto la tesi per cui questi investimenti siano legati unicamente all'utenza. Questo, infatti, è un gatto che si morde la coda: coda: probabilmente nel Sud c'è meno utenza perché ci sono meno infrastrutture, perché i treni funzionano peggio, perché c'è molto più binario unico che altrove, anche in alcune tratte dove ciò non è storicamente giustificabile. A questo proposito io credo che noi avremmo il dovere di porre all'ordine del giorno due questioni e prendo il suo intervento solo come l'anticipazione di comunicazioni molto più corpose. Si tratta di due questioni che emergono in tutta la loro portata strategica ed epocale

l'organo irresponsabile, anche dal punto di vista economico, delle origini (della legge n. 281 del 1970), ma non ha trovato ancora una sua definizione di autonomia e dunque di responsabilità. E questo dato viene tragicamente alla luce da quanto lei ci ha riferito e dal tentativo di trovare degli accordi che non sono affatto scontati. Dall'altra parte, vi è la questione del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno. Chiunque prenda un treno da Roma in giù si rende conto che quella è la metafora di una questione più grande, di un divario tra il Nord e il Sud che è tornato a crescere,

spalle di quelle parti del Paese che sono più sviluppate. Il nostro Mezzogiorno produce più del 30 per cento del PIL nazionale, non il 3 per cento come la Corsica rispetto alla Francia: non possiamo trattarlo allo stesso modo. Devo dire che che ho visto le conclusioni dei primi tavoli tra il Governo e le Regioni e gli obiettivi che si sono dati; è veramente difficile, anche con la buona volontà, rintracciare una strategia. Negli anni passati vi sono stati grandi dibattiti sulla questione meridionale, sulla necessità di lasciarla allo spontaneismo dei territori e delle Regioni oppure di avere una strategia di tipo centralistico. Quelle opzioni potevano forse essere un po' ideologiche, ma erano opzioni e linee di sviluppo; oggi non c'è niente. Non si può dire che la nostra politica meridionale sia una cattiva politica, perché in realtà una politica non c'è. Se quanto avvenuto - al di fuori delle polemiche - ci porterà a porre all'ordine del giorno questo problema come problema nazionale e come problema di coesione nazionale, forse quello sarà il modo migliore per onorare le vittime innocenti che ieri hanno hanno perso la vita anche per un'arretratezza lontana. Quel popolo delle formiche, che è stato schiacciato da qualcosa di più grande, potrà tornare ad essere un popolo fiero, laborioso e pacificato perché ha avuto le risposte che si aspettava di avere. non ci sono parole sufficienti per descrivere la tristezza e il dolore suscitati da una tragedia di proporzioni immani, come quella avvenuta ieri tra Andria e Corato. Mai avremmo potuto pensare, nel 2016, in un'era di sviluppo straordinario sul piano delle tecnologie e delle comunicazioni, di doverci trovare a dibattere di uno scontro tra treni, di dover fare i conti con una situazione impressionante, per cui, nella zona dell'incidente, è stato addirittura necessario montare un vero e proprio ospedale da campo. Eppure è successo e noi qui, oggi, ci troviamo a rendere un omaggio commosso alle vittime e a stringerci intorno al dolore lancinante dei loro cari. E qui, colleghi, desidero evidenziare che non è il tempo né delle polemiche né delle strumentalizzazioni. Certo, nei prossimi giorni e a mente più fredda, potremo e dovremo approfondire temi che sono stati riportati alla luce anche sulla stampa dal disastro di ieri, a partire dal mancato raddoppio - pure previsto e finanziato da molti anni - della tratta ferroviaria in questione e dalla mancanza di qualsiasi sistema di sicurezza lungo la stessa. Peraltro, siamo certi che le istituzioni preposte faranno tutto quanto nelle loro possibilità per capire cosa è successo e perché. È assolutamente necessario chiarire nel minor tempo possibile le cause e, quindi, la dinamica dell'incidente. Viste le proporzioni disastrose della tragedia, sarà un lavoro certamente complesso, ma che necessariamente dovrà portare a risposte chiare: lo si deve alla memoria delle vittime, così come ai loro familiari, ma anche, colleghi, all'intero Paese che ha assistito sgomento, con sconcerto e partecipazione a quanto accaduto. Ma ora, ripeto, è il tempo del dolore e della preghiera, oltre che della solidarietà, che desidero indirizzare ai familiari delle vittime, anche a nome del Gruppo parlamentare AL-A. A proposito di solidarietà, ritengo di assoluta importanza condividere una riflessione su questo Paese che - mi sento di dirlo senza retorica - ha seguito con apprensione e reale partecipazione quanto accaduto. accaduto. Spesso, a volte con ragione, anche come specchio delle tensioni esasperate che si registrano nelle Aule parlamentari, consideriamo il Paese diviso al suo interno e non sufficientemente solidale nell'epoca odierna segnata dalla globalizzazione e da tensioni sociali ed economiche di portata epocale, ma nei momenti di difficoltà e dolore quello stesso Paese mostra un volto umano e solidale di straordinario spessore. Desidero fare un riferimento particolare alla generosità e al calore dimostrati dalla moltitudine di cittadini pugliesi residenti nei territori del barese e del Nord barese che si sono recati nelle strutture ospedaliere, dando una risposta straordinaria alle richieste in tal senso, ma anche in molti casi anticipandole, per donare il loro sangue a fronte dell'emergenza verificatasi. Ho trovato commoventi le dichiarazioni di alcuni dei moltissimi studenti di medicina che, trovandosi lì per studiare, hanno fatto la fila al Policlinico di Bari.

Sono questi i valori di solidarietà e fratellanza che in tante occasioni hanno consentito al nostro Paese di affrontare momenti di estremo dolore e di assoluta difficoltà. valori, peraltro, ho ritrovato anche nel lavoro indefesso delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dei volontari, della Protezione civile e degli operatori sanitari, protagonisti di un impegno smisurato tra le lamiere dei treni. L'autentica gara di solidarietà e generosità di ieri nelle strutture sanitarie ne è un esempio commovente. Signor Ministro, esprimo apprezzamento per la rapidità con la quale sia lei che il Presidente dei Consiglio vi siete recati ieri stesso sul luogo del disastro, così come per le vostre parole, misurate e attente, volte a comunicare da una parte la vicinanza del Governo e dall'altra il rispetto totale per il lavoro della magistratura e di tutti gli organi preposti a fare luce. Quanto avvenuto - in conclusione, rivolgo al Governo, nell'ambito dei suoi compiti, questa breve riflessione - deve farci comprendere come ancora molto debba essere fatto per la sicurezza delle infrastrutture in molte parti del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno che registra purtroppo ancora oggi *gap* insopportabili. Che tragedie come questa non si ripetano più!

La situazione di fatto è questa: una linea a binario unico, una linea elettrificata, materiale rotabile nuovo, tratta senza particolari complessità geomorfologiche, però linea a bassa frequenza di movimento (almeno queste sono le informazioni che ho). Si è però previsto il raddoppio della linea con stanziamenti anche importanti in anni ancora lontani. la differenza di normativa tra la gestione delle linee nazionali e quelle locali e la possibilità di intervenire in momenti momenti lontani allorquando si è fatta l'elettrificazione. Ho fatto il riepilogo di questa situazione, perché di certo la responsabilità del Governo attuale non esiste e sono anzi apprezzabili e apprezzati l'intervento tempestivo e la sensibilità mostrata rispetto ai territori, alle ai territori, alle famiglie e a tutti coloro che sono stati coinvolti nella tragica vicenda che abbiamo di fronte. È anche probabile che l'accaduto sia frutto di un errore umano, dovuto all'assenza di sistemi di segnalamento e di sicurezza moderni e adeguati: questo è il punto. In passato si è scelto il raddoppio costoso, invece di mettere la linea subito in sicurezza.

ma non stanziamenti razionali. Perché per quel territorio, prima di avere il raddoppio, trattandosi di linea a bassa frequenza e a bassa difficoltà geomorfologica, sarebbe bastato un sistema di segnalamento adeguato. Il collega Quagliariello ha richiamato la presenza nel nostro Paese e anche in quei territori di competenze professionali e imprenditoriali di primaria importanza mondiale. È vero: l'Italia è all'avanguardia nel sistema del controllo ferroviario e della produzione di sistemi ferroviari. però pensato che quel territorio avesse bisogno del raddoppio, perché era importante portare in quel territorio 100 o 150 milioni di euro,

la corsa agli stanziamenti importanti, per fare i raddoppi e le opere, da "appendere sul petto come decorazioni" per chi svolge attività parlamentare. di avere la guida di un'azienda importante del Nord, che svolgeva attività nel settore delle gomme e ferroviario, la SATTI di Torino, oggi azienda nell'effettuare importanti investimenti nel settore ferroviario ci siamo posti due problemi: quello del materiale rotabile e quello della sicurezza sulla linea. Certo, anche l'elettrificazione è un elemento importante, ma insieme all'elettrificazione, colleghi, la realizzazione di un sistema di controllo e di segnalamento adeguato e all'altezza della situazione si può attuare con risorse molto limitate. Il collega Borioli, che è stato assessore ai trasporti della Regione Piemonte, sa cosa voglio dire. Dunque, la responsabilità è certamente nel fato e potrà essere ricercata dalla magistratura, che lo farà, ma credo che la responsabilità stia anche nelle nostre scelte, che spesso sono dettate da interessi di carattere

ma voglio ricordarlo anche qui: come senatori siamo parlamentari della Repubblica italiana e non di un pezzo di un territorio piuttosto che di un altro. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, oggi anche in quest'Aula sono ricorrenti parole come «dolore», «strazio», «profondo cordoglio»; confesso però, al di fuori di ogni ritualità, che sono i sentimenti che da ieri mattina mi stringono come un nodo alla gola e mi investono, non solo come senatore della Repubblica e come cittadino italiano, ma soprattutto - lo comprenderete - come pugliese. Da ieri si susseguono nella mente le immagini di quelle lamiere diventate briciole, di quei volti del dolore che dalle campagne pugliesi hanno raggiunto l'Italia intera, ma anche degli uomini e delle donne a me vicine, amiche o solo conoscenti, che percorrono giornalmente quel tratto di strada, quel pezzo di 70 chilometri di ferrovia ancora una volta macchiata di sangue di sangue e dolore, un dolore che io credo ingiusto e inaccettabile. Davanti a questa tragedia il primo imperativo categorico deve essere la necessità di non dare vita a inopportuni esercizi di sciacallaggio politico in ogni direzione sia dal centro verso la periferia - le Regioni - sia in senso contrario. Allo stesso modo, ci corre l'obbligo di non vestire questo terribile incidente come un'ignobile occasione per sistemare conti di natura politica. È il momento di superare la narrazione che solitamente si innesta sul limitare di queste tragedie; una narrazione che diventa, soprattutto nel nostro Mezzogiorno, caro collega Buemi, quasi un incantesimo maledetto, perché, superata l'emergenza, tutto ritorna dannatamente come prima, o almeno quasi tutto, se pensiamo a chi rimarrà con il dolore straziante della perdita di un proprio caro. Rincuorano - non sembri superfluo che lo rimarchi anche io - la pronta risposta della macchina dei soccorsi, la grande solidarietà del popolo italiano e la generosità dei pugliesi; ma non basta: occorre che ciò sia da monito ad agire con solerzia e oculatezza. Ringrazio sinceramente, quindi, il ministro Delrio per la relazione puntuale e misurata sul tragico evento di ieri,

Signor Ministro, oggi, secondo me, da quest'Assemblea e dal Parlamento italiano, ma - soprattutto - dalla polvere di quella terra rossa, arsa e riarsa dal sole cocente delle campagne di Andria e Corato, deve emergere la volontà di agganciare finalmente e definitivamente l'innovazione nel sistema delle infrastrutture per tutto il nostro Paese: tutto e non solo di un pezzo. L'Italia è divisa in due, caro collega Buemi. Cari colleghi, non ci sono sofismi e tantomeno sofisti in grado di azzardarsi ad affermare e sostenere il contrario. non è divisa in due parti per mera responsabilità del popolo del Sud o di chi lo amministra. Guardiamo alla realtà con la lealtà che si deve ad un'intera comunità che si interroga. Essere leali significa, ad esempio, non indugiare sulle cifre.

Caro collega Buemi, caro collega della Lega Nord, questi sono i numeri. In poche parole, quello che si spende per quadruplicare il solo tratto che collega Lucca a Pistoia è pari a tutta la spesa che spetta all'intero Mezzogiorno. Insisto solo per continuare a dar forma a questa mostruosità: in tutto il Sud i treni pendolari sono meno di quelli della sola Lombardia. Come se non bastasse, stretti nella tenaglia di mancati investimenti nelle infrastrutture, tutto quello che rimane viene ulteriormente spolpato e aggredito dalla politica di riduzione dei costi - la cosiddetta *spending review* operata sia dal pubblico che dal privato spesso nella direzione peggiore, quella che morde sulla carne viva delle persone, dei più deboli. Il trasporto pubblico locale morde lì. L'elemento che oggi emerge da quelle lamiere sbriciolate, allora, è che sulla tratta Bari Nord non era ancora attivo un sistema di segnalazione dei binari occupati, ossia un sistema di sicurezza che blocchi il treno in caso di ingombro sui binari. Binari, questi, interessati negli ultimi decenni da numerosi incidenti (più di 120 incidenti negli ultimi quindici anni) e da altrettante, troppe vittime, che hanno accompagnato l'esistenza di quel pezzo di infrastruttura ferroviaria. Numeri che restituiscono di fatto la certezza che quanto avvenuto ieri sul quel tratto di ferrovia pugliese non può essere inquadrato esclusivamente nella fattispecie dell'errore umano. Signor Ministro, colleghi, nella doverosa ricerca dell'errore umano, dobbiamo avere il coraggio di non limitare il nostro sguardo al dito, ma dobbiamo obbligatoriamente mirare alla luna. luna. Attribuire per intero la colpa al fonogramma o al mancato fonogramma, ad una telefonata fatta o mancata, ad una sbagliata interpretazione del "via libera" da parte di uno dei macchinisti o di tutti e due significa non comprendere e continuare ad ignorare, ancora nel 2016, che in alcune parti dell'Italia non si è operato opportunamente per applicare ovvi e già operanti sistemi che riducono l'errore umano, riducono il rischio e aumentano la sicurezza. Non possiamo ricercare la distrazione del macchinista se continuiamo ad ignorare quella del legislatore, e quindi anche nostra, nell'affrontare la questione dell'inadeguatezza delle infrastrutture in alcune Regioni del nostro Paese. È un problema vero di coesione. Studenti e lavoratori - tutti pendolari - ci raccontano di una condizione delle ferrovie regionali e locali insopportabile. E in questo momento il mio pensiero torna alle Ferrovie del Sud-Est, che ci narrano un racconto di sprechi e di scandali al quale io spero questo Governo voglia finalmente porre rimedio, che non è solo un freno, ma una dannata zavorra per lo sviluppo di queste terre, un vergognoso disagio a cui in casi come questo si aggiunge anche l'aggravante di rischio. Concludo questo Presidente, chiedendo ed invocando un intervento straordinario da parte del Governo e un impegno immediato da parte delle istituzioni competenti. Altrimenti si rischia veramente di fare anche questa volta oltraggio alle vittime e di continuare a perpetrare tale delitto nei confronti di un intero territorio e di un'intera comunità che si interroga.

ci stringiamo con grande afflato di solidarietà alle famiglie delle vittime. Lo abbiamo fatto e lo abbiamo ripetuto; queste espressioni di solidarietà non sono mai troppe, in questo momento di dolore, per le famiglie pugliesi. Ci accodiamo e ci uniamo al coro di apprezzamenti e di elogi per come ha funzionato la macchina della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e della solidarietà tutta, che il popolo pugliese orgogliosamente ha saputo mettere in moto. Apprendiamo però con stupore e con allarme dalla sua relazione alcune note che chiaramente ci sorprendono. Mi riferisco al sistema di sicurezza sul binario unico con il blocco telefonico; chiaramente

di sistemi di sicurezza, che secondo me dovrebbero essere ormai abbondantemente superati. Quindi mi rendo conto che, se c'è ancora il blocco telefonico nella linea oggetto dell'odierna tragedia, mancano gli appositi

ho saputo che la sicurezza di esercizio su tutte le linee ferroviarie del Paese, che non sono di competenza della RFI, fra cui la Ferrotranviaria SpA o la Circumetnea, purtroppo non risulta affidata all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Pertanto non vengono garantiti al viaggiatore i migliori ed adeguati *standard* internazionali di sicurezza ferroviaria e le opportune tecnologie all'avanguardia nel settore. Dunque, viene purtroppo trascurato il servizio pendolari e quello turistico cui tali linee sono vocate. Signor Ministro, per evitare altre possibili sciagure ed assicurare la migliore prevenzione del rischio, occorre garantire certamente la migliore sicurezza, affidabilità ed efficienza di tutte le linee ferroviarie, soprattutto di quelle regionali al servizio dei pendolari e del turismo, che finora non sono state sottoposte, da quello che apprendo, ai rigorosi *standard* internazionali e alla rigida ed efficace vigilanza e controllo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Quindi, se è vero che il binario unico - lei ha richiamato l'incidente in Germania - che si ritrova in oltre la metà della rete ferroviaria gestita dalla RFI non è in quanto tale la causa di carente sicurezza, bisogna chiedersi perché la tecnologia, che accorre in maniera decisiva e quasi matematica in caso di inefficienze umane, sia obbligatoria e operativa solamente sulla parte gestita direttamente dalla RFI e non su quella data in concessione. Evidentemente dobbiamo anche rivedere le convenzioni ed i contratti di concessione con le società private. Il Governo, a parer mio, si deve quindi attivare perché il controllo operativo di questa parte di rete ferroviaria, considerata secondaria passi alle dirette competenze (competenze non di gestione, chiaramente) e al controllo della sicurezza della RFI, al fine di rendere omogeneo il grado di sicurezza in tutto il Paese ed assicurare, nel contempo, mirati investimenti in tecnologia ed adeguati miglioramenti dei livelli Il disastro di ieri, mi consenta, signor Presidente, può però fornire lo spunto per un ragionamento più ampio, perché è stato detto da molti colleghi

tratte a binario unico (1.200 chilometri) e tratte a doppio binario (soltanto 180 chilometri). La ferrovia Palermo-Messina, che è stata oggetto di mie numerose interrogazioni (purtroppo senza risposta),

Manca su questa tratta anche una progettazione di tipo preliminare ed una pianificazione. Pertanto, la invito, signor Ministro, così come ho fatto anche ai tempi del ministro Lupi e come continuerò a fare, a provvedere perché si possa dotarci di possa dotarci di un progetto preliminare da inserire nella programmazione. Mi richiamo all'intervento del senatore Buemi, perché è vero che da parte degli enti locali e delle Province a volte le segnalazioni non sono sufficienti, perché si chiedono cose che probabilmente servono meno di quelle di cui c'è effettivamente bisogno. Signor Ministro, la invito anche a guardare attentamente il Piano per il Sud, perché tutte le richieste progettuali e la pianificazione che arrivano da questo programma probabilmente non saranno utili per poter colmare le debolezze infrastrutturali, che invece sono importanti. I soldi del Piano per il Sud non servono a fare la riqualificazione urbana o a mettere una coccarda sul petto di un sindaco, ma servono anche a rimediare

è che le nostre istituzioni, a tutti i livelli e con il dovuto grado di coordinamento anche con gli operatori privati, devono imparare a programmare, progettare e spendere le risorse, che in molti casi pure ci sono, per il trasporto regionale e locale. Una dotazione infrastrutturale, tecnologicamente avanzata nel settore ferroviario dell'intero Paese, innesca un circolo virtuoso verso lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione e, allo stesso tempo, può ridurre drasticamente le possibilità che la nostra società sia sconvolta da una tragedia come quella che avant'ieri ha colpito la comunità pugliese e l'Italia tutta.

prima di tutto esprimiamo vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite, ma ringraziamo anche i soccorritori e i donatori di sangue, che così celermente hanno operato per ridurre al minimo le conseguenze Questo, però, sicuramente non è da considerare un incidente. Vi sono delle negligenze che non devono essere ricercate nel personale,

salvaguardate dalla possibilità dell'incidente derivante dal fattore umano. Il personale è vittima anch'esso di questa tragedia. Ora non è tempo di fare polemiche e quindi non voglio dilungarmi sulla quantità di soldi stanziati al Nord piuttosto che al Sud o per l'alta velocità piuttosto che per il colore delle vetture piuttosto che per il condizionatore d'aria: adesso è tempo di andare più nel concreto, di andare a vedere quali sono le soluzioni possibili per evitare che questi incidenti

più appropriatamente consenso telefonico, perché non si tratta di un blocco a tutti gli effetti. Quindi, il consenso telefonico lascia la possibilità di errore e di

Come è stato giustamente detto, la colpa non è del binario unico, perché sul binario unico si può tranquillamente intervenire con sistemi di sicurezza che appropriatamente evitano queste possibilità di incidentalità.

ai convogli di passare senza che vi siano interferenze tra di loro. Altro problema sono le linee in concessione, perché attualmente le linee in concessione derivano non dagli uffici nazionali dell'ANSF, quindi non dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ma dall'USTIF, dall'ufficio speciale trasporti a impianti fissi. Questo implica, comunque, una certa libertà, anche per le Regioni, di scegliere lo *standard*

Le linee FS non hanno questo tipo di blocco, di consenso telefonico, che è stato eliminato parecchi anni fa. Quindi, questo è uno dei motivi per cui noi siamo per l'infrastruttura pubblica. Poi, il gestore può essere privato, eventualmente, ma con delle regole d'ingaggio, come è stato detto altre volte, ben specificate. La sicurezza deve essere prioritaria su qualsiasi cosa.

noi vorremmo un censimento delle linee che effettivamente sono in questo stato o in stati similari e quindi avere contezza di queste situazioni critiche.

affinché queste cose non succedano più e gli *standard* di sicurezza passino interamente in carico all'ANSF. Questo implicherebbe l'introduzione di blocchi a salvaguardia dei tracciati. Arrivo alla alla terza proposta: visto e considerato che i tempi comunque sarebbero troppo lunghi per l'installazione di blocchi normali (a cavo, con cavi di relazione, garitte e quant'altro),

in Lombardia è in sperimentazione un ERTMS di livello 2 sulle linee tradizionali: è il blocco radio, tanto per intenderci. Il blocco radio sarebbe di facile introduzione, molto più veloce e sicuramente a minori costi di installazione. Sarebbe subito operativo ed è quello che chiediamo adesso. Se vogliamo veramente fare qualcosa per i cittadini, perché non succedano più incidenti di questo tipo, bisogna operare da subito e bisogna che quei soldi che voi chiamate la "cura del ferro" - non voglio fare polemiche - siano da subito spesi in salvaguardia e sicurezza, perché questo deve essere fatto. Non si può parlare di nient'altro se non di sicurezza. Arrivo da vent'anni di lavoro nel campo del segnalamento ferroviario e posso assicurarvi che il segnalamento ferroviario italiano è un fiore all'occhiello un motivo di vanto per gli operatori ferroviari italiani. Non facciamo che diventi il nostro tallone di Achille.

la ringrazio per aver accolto prontamente l'invito rivoltole da più parti, ivi compresa la Commissione lavori pubblici e comunicazioni che mi onoro di presiedere, a svolgere un'informativa sul disastro ferroviario. Al di là dell'appartenenza politica di ciascuno di noi, credo che bisogna dare atto a lei di essere tempestivamente intervenuto sul luogo della sciagura e per questo, a nome del Gruppo di Forza Italia, la ringrazio. Comprendo perfettamente che non sarebbe stato possibile dopo ventiquattr'ore potere disporre con esattezza di tutte le informazioni sull'incidente, né soprattutto avere contezza delle cause che hanno determinato questo tragico scontro frontale tra due convogli. Ma anche dalle sue parole si evince che qualcosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza. Arrivare a fare totale chiarezza è quindi doveroso per le vittime, per i loro familiari e per far sì che tali accadimenti si possano evitare in futuro. Non ho dubbi che la verità sarà acclarata, ma, anche per l'esperienza che ho potuto maturare sul campo, mi permetto di consigliarle di stare all'erta, di controllare con la massima attenzione l'evolversi delle indagini stimolando gli investigatori a fare presto e se possibile bene. Oggi aprendo i giornali, però, ho avuto una sorpresa: sembrerebbe che l'unico colpevole del disastro sia il binario unico. Si privilegia purtroppo, anche in questa tragica circostanza, il sensazionalismo, la ricerca immediata di un colpevole e lo si trova in modo del tutto arbitrario e incredibile per offrirlo velocemente all'opinione pubblica. Stavolta è il turno del binario unico e, ovviamente, di tutta la classe politica del Paese, incapace per non aver saputo spendere oculatamente i soldi pubblici, non realizzando il doppio binario in tutta Italia e una rete ferrata moderna. È assurdo. Sappiamo tutti che in Italia oltre il 60 per cento della linea ferroviaria è a binario unico, in linea con l'Europa: anche in Europa è così. è allora la realtà infrastrutturale ferroviaria e se davvero il colpevole fosse il binario unico, di tragedie come questa pugliese se ne dovrebbero contare a centinaia. Per fortuna non è non è così perché, come ci spiegano i tecnici del ramo, binario unico non è sinonimo di insicurezza. Il doppio binario non offre maggiori garanzie di sicurezza - lo ha detto molto bene anche lei - ma maggiore capacità di traffico ferroviario. per cento della rete gestita dalla RFI sono installati, infatti, i più moderni sistemi di sicurezza che riescono a impedire incidenti come quello accaduto in Puglia. Ci sono, invece, brevi tratti di rete regionale che non hanno ancora installato sistemi moderni di sicurezza e che operano con meccanismi antidiluviani, come l'uso del telefono, con cui comunicano capistazione e macchinisti. A quanto pare - e lo ha confermato oggi - la tratta dove è accaduto il disastro ricade in quest'ultimo caso ed è evidente che qualcosa non abbia funzionato nella comunicazione tra macchinisti e capistazione. Oggi ogni sforzo deve preliminarmente essere diretto a scoprire cosa e perché non abbia funzionato, ancor prima di risalire a eventuali responsabilità personali di qualche addetto. Dico una banalità, ma è evidente che su quel binario c'era un treno di troppo: su questo non ci sono dubbi. Assumere il disastro della Ferrotramviaria di Bari per gettare la croce addosso alla politica, alle sue inefficienze, ai suoi sprechi mi pare improprio e demagogico. Questo - voglio dirlo con chiarezza - non significa assolvere tutto e tutti o scaricare responsabilità. Voglio semplicemente dire che, di fronte ad un disastro

per il recupero della politica nel nostro Paese. Credo quindi che occorra intensificare da subito l'attenzione e lo sforzo finanziario per tappare le falle nei sistemi di sicurezza, adeguandoli nei tempi più rapidi alle più moderne tecnologie, e di pari passo cercare in ogni modo di ammodernare la rete ferroviaria secondaria che, specie in alcune aree del Meridione, risulta fatiscente e inadeguata. Signor Ministro, lei oggi ha voluto sottolineare che il Governo di cui fa parte ha invertito la tendenza del passato. Vede, signor Ministro, del numero di stanziamenti di risorse sulla carta, che spesso si spostano da un capitolo all'altro, o che vengono recuperate perché non spese prima, o che all'ultimo momento vengono dirottate su altre dirottate su altre scelte magari a causa di emergenze di ogni tipo, di finanziamenti che non si tramutano in vere realizzazioni, si potrebbero scrivere tanti volumi. Ciononostante, qualora l'inversione di tendenza cui lei ha fatto riferimento dovesse realmente essere coronata da fatti tangibili, ossia da realizzazioni infrastrutturali, noi gliene daremo volentieri atto perché riteniamo, da forza di Governo quale siamo stati e vogliamo tornare ad essere, che il Paese e l'interesse dei cittadini vengano prima di tutto. Detto questo e ritornando al binario unico (mi scuso se insisto, ma la lettura dei giornali di questa mattina mi ha innervosito), far credere in maniera semplicistica che era possibile e necessario realizzare il doppio binario dappertutto, la trovo una *boutade* che serve solo a fare confusione, gettare discredito e allarmare i cittadini. confermare al Ministro e al Governo che la Commissione che presiedo è pronta a offrire ogni contributo, come ha sempre fatto in questi anni. Desidero infine - ma non infine e chiedo scusa se ho usato questo termine, improprio per quello che sto per dire - far giungere il cordoglio del Gruppo Forza Italia ai familiari delle vittime così duramente colpiti, un augurio di pronta guarigione ai feriti e un grazie ai soccorritori che ancora una volta svolgono con impegno e grande professionalità

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei iniziare dal racconto del dolore provato nell'apprendere del tragico incidente ferroviario, ma è veramente difficile dire cosa si prova nel vedere tante vite spezzate in un giorno normale, come tanti, mentre non temevano nulla perché facevano quel tratto ogni giorno, magari da tanti anni. Allora mi posso limitare ad esprimere la vicinanza autentica mia e del mio Gruppo a tutti i parenti delle vittime e a tutti i feriti, insieme alla promessa di fare in modo che l'accertamento della verità sulle cause sia rapido ed approfondito. Emergeranno nei prossimi giorni le storie ed i volti delle troppe vittime di questa tragedia; per tutti noi saranno storie e volti che ci torneranno in mente, fino a tormentarci, ogni volta che saremo chiamati a lavorare per migliorare il sistema di trasporto ferroviario nel nostro Paese. E questa non è una promessa ma una garanzia. Il nostro Presidente della Repubblica l'ha giustamente definito un disastro inammissibile, e infatti lo è. È una cosa che non doveva avvenire e per la quale non ci si può, e non ci si deve, rassegnare ad ipotesi di fatalità. Stare però qui, in quest'Aula, a cercare di definire da lontano le responsabilità sarebbe un atto sbagliato; quanto ora ci compete è cercare di capire cosa possiamo fare di più e di meglio per evitare che tragedie simili possano ripetersi. Sappiamo che il trasporto ferroviario dei pendolari è un sistema da tempo in difficoltà in tutto il nostro territorio, perché è stato trascurato per molto tempo e perché continua a non essere considerato remunerativo.

Per cui non siamo di fronte ad una incapacità strutturale o ad una storia di Sud arretrato; siamo, più probabilmente, di fronte ad una serie di cause che, messe insieme, hanno generato il rischio e, purtroppo, la tragedia. Cause strutturali, come la mancanza del doppio binario (che pure era stato finanziato da tempo e il relativo appalto era proprio in via di assegnazione) e soprattutto la sicurezza, affidata ancora solo alle comunicazioni telefoniche, e forse cause umane, che saranno sicuramente attentamente vagliate. Sentimenti contrastanti sono stati vissuti dall'intero Paese per tutta la giornata di ieri. Del resto, una tragedia di proporzioni impressionanti come quella avvenuta suscita istintivamente apprensione e dolore, ma anche rabbia e sgomento. Suscita anche intransigenza per sapere la verità, per acclarare responsabilità e conseguentemente pretendere giustizia. Ma anche sentimenti di autentica commozione cui aggrapparsi per continuare a sperare nella vita e volere, questa volta davvero, che non si ripeta mai più. Commozione è stata suscitata dalle tante lacrime viste versare, ma ancor di più dai silenzi e dallo stupore degli occhi smarriti di chi non si può capacitare. In quest'Aula, come molti che mi hanno preceduto, voglio ringraziare a nome del mio Gruppo tutti coloro che da subito hanno lavorato incessantemente per soccorrere le vittime: i volontari, i medici ed i paramedici, gli appartenenti alle varie forze di polizia, la prefettura che ha collaborato con il sistema di Protezione civile. Un impegno straziante che va avanti ancora adesso. Grande commozione ho provato anche per le migliaia di cittadini comuni che spontaneamente si sono riversati negli ospedali, per fare il gesto più spontaneo e più utile: donare il sangue per soddisfare il fabbisogno necessario. Più di altre volte è apparsa un'Italia che, nell'inammissibilità della tragedia, ha dato l'impressione di sapere cosa si deve fare in queste circostanze. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto ed era pronta per l'uso. La cultura della protezione civile è cresciuta in questi anni grazie al lavoro di educazione diffuso, a partire dalle scuole come prima sensibilizzazione, e alle periodiche esercitazioni che servizi dello Stato e associazioni di volontariato realizzano per migliorare l'integrazione delle proprie prestazioni. In questo contesto, credo che tutti possano concordare sul fatto che anche lei, signor Ministro, e il Presidente del Consiglio avete fatto il vostro dovere.

che non c'è stata nessuna espressione di vivo entusiasmo per gli investimenti in corso da parte del Ministro, ma la consapevolezza di attivare da subito tutte le risorse disponibili per comprendere bene cosa sia successo, assicurando ai parenti ed ai sopravvissuti tutto il sostegno necessario, con la piena collaborazione della Regione e dei Comuni della zona. Eppure, anche in questi momenti difficili abbiamo l'obbligo di guardare avanti. Guardare avanti deve voler dire che gli investimenti sulla sicurezza in sistemi automatici di protezione non possono prevedere eccezione alcuna, sia che riguardino tratte delle Ferrovie dello Stato sia, ancor più, che si tratti di ferrovie concesse. Essere un Paese normale significa non fare distinzione di priorità in termini di sicurezza tra servizi a mercato e servizi universali, tra tratte regionali e linee ad alta velocità. Certo il dolore richiama alla memoria il disastro di Crevalcore e la tragedia sconvolgente di Viareggio, pur sapendo che si tratta di fattispecie tra loro differenti. Ma se la memoria va spontaneamente a queste tragedie è perché i trasporti collettivi di massa, usati in prevalenza da studenti e lavoratori, non possono consentire approssimazioni o atteggiamenti indulgenti. Vorrei far notare al senatore Quagliariello che già sono state attivate Commissioni di inchiesta previste dai diversi livelli istituzionali. Mi sento di affermare che di queste il Parlamento pretenderà

per assumere, se necessario, come credo, i provvedimenti legislativi che si renderanno più opportuni. Imparare dalle tragedie è l'unica risposta seria che possiamo dare per fare in modo di non dover più piangere per morti inammissibili.

Onorevoli colleghi, le Commissione riunite affari esteri e difesa non hanno concluso l'esame della legge quadro sulle missioni internazionali all'ordine del giorno.

Signor Presidente, troppo spesso accade che in Italia ci troviamo ad affrontare questioni che riguardano il non rispetto del paesaggio e dell'ambiente, cosa che sta avvenendo in queste ore ad Ostuni, splendida cittadina pugliese, luogo turistico e di mare, dove si sta realizzando una vasca di raccolta liquami. Il problema, in questo caso, è dove la si vuole realizzare. Presidente, la vasca di liquami la stanno costruendo su una spiaggia libera di una località che si chiama Pilone; sì, proprio sulla spiaggia a ridosso del mare, area fra l'altro soggetta a vincoli paesaggistici. Si tratta di un'area protetta a forte valenza turistica ed esattamente di fronte o, meglio ancora, a pochissimi metri da una torre saracena La popolazione, amministrazione locale compresa, è insorta contro questa scellerata decisione e - badate bene - non contro la realizzazione della vasca, che va fatta, ma sulla scelta del luogo. Viene così proposto dal Consorzio Villaggio Torre San Leonardo di Pilone un progetto alternativo che prevede la stessa opera, ma a 300 metri verso l'interno, lontano dalla spiaggia e dal mare, luogo fra l'altro previsto nel progetto originario risalente al 2005 e che era divenuto anche progetto esecutivo ma poi mai realizzato.

Ebbene, dalla documentazione tecnica fornita dal comitato, dai cittadini e dal sindaco non sussiste alcuna pendenza tale da pregiudicare l'opera. Inoltre, ho effettuato personalmente un sopralluogo e ho verificato esattamente questo,

Vista la ferma opposizione della popolazione, il presidente della Regione Puglia, Emiliano, circa quattro mesi aveva fa promesso una nuova conferenza dei servizi al fine di comparare i due progetti, ma sembra che abbia fatto marcia indietro, rimangiandosi la parola data. dunque estremamente grave non solo la realizzazione di questa vasca in un luogo non idoneo e a rischio ambientale, ma trovo anche grave che Emiliano prenda in giro i cittadini pugliesi.

permettendo ai cittadini tutti di partecipare a una decisione tanto importante.